Signor Presidente, la ringrazio veramente per avermi dato la parola a nome mio personale e del senatore Vimercati, ma anche a nome della mia città, Sesto San Giovanni, che si è sentita profondamente offesa dalle parole che il senatore Gasparri ha pronunciato in quest'Aula lo scorso venerdì e che sono state riprese da molte televisioni. Le sue parole sono suonate come una condanna senza appello. Ha definito Sesto come una città dove di padre in figlio i sindaci alimentano un sistema di illegalità

abbia in un certo senso conservato - io posso dirlo - un certo livore ideologico, forse alimentato dal nome con cui viene definita la mia città, ex Stalingrado. Ma penso che, dalla caduta del muro di Berlino ad oggi, molta acqua sia passata sotto i ponti, e il soprannome che questa città conserva, nonostante i tanti cambiamenti politici, economici e sociali, a sottolineare soprattutto la sua capacità di lotta, prima contro il fascismo, poi nella Resistenza - e da lì il suo riconoscimento a città medaglia d'oro al valore militare - e successivamente nelle lotte per la conquista dei diritti del movimento operaio e del movimento delle donne. Gasparri, la resistenza eroica, anche negli scioperi del '43, a fronte della minaccia di rappresaglie del generale tedesco Zimmerman, costò la deportazione, la tortura e la fucilazione di tanti lavoratori sestesi. Sesto poi nel dopoguerra, dopo aver salvato le sue fabbriche, ha saputo affrontare con spirito solidale il raddoppio della popolazione immigrata dal Sud povero del Paese e ha saputo opporsi con tutte le sue forze al terrorismo nero e poi a quello rosso, che hanno insanguinato gli anni '70 e '80. Negli anni '80 e '90 abbiamo perso 22.000 posti di lavoro, ma le lotte per la difesa del posto di lavoro e per costruire un futuro per la città sono state affrontate con grande dignità, compostezza e spirito costruttivo. Non ci sono stati né progetti speciali né finanziamenti speciali per affrontare la riconversione di oltre 2 milioni di metri quadri di aree industriali dismesse, rischiavano di essere un buco nero che poteva ingoiare la città. Per questo, presidente Gasparri, anche suoi amici del PdL di Sesto San Giovanni hanno chiesto che l'attuale amministrazione vada avanti per approvare il piano territoriale nel settembre prossimo. Sanno anche loro qual è la posta in gioco. Nessuno di noi vuole fare sconti a qualcuno, se ci saranno responsabilità. Ma questo non può voler dire trascinare nel fango una città

Signor Presidente, potrei rispondere alla lagnanza della senatrice Bassoli ricordandole la libertà di espressione e, ancor più, l'insindacabilità dei giudizi espressi nelle Aule parlamentari. Se anche questi dovessero cadere sotto la scure della censura, o peggio sotto il vaglio della magistratura, verrebbe meno un'ulteriore residua garanzia che dà un senso al nostro ruolo di rappresentanti del popolo. E a perdere sarebbero, ancora una volta, il Parlamento tutto e le ragioni della persistenza di una sua centralità. Ma non è solo questo in discussione, e vorrei brevemente ricostruire i fatti. Durante la discussione del provvedimento sulla parità fra le parti nel processo, in un accorato intervento subito dopo la decisione di porre la fiducia, il collega Zanda ha detto in quest'Aula che ci trovavamo a un passo dal regime. E poiché i regimi vi sono quando l'opposizione non ha strumenti per opporsi alla tirannia della maggioranza e la maggioranza non ha da temere quel fisiologico ricambio su cui si basa la democrazia, il senatore Zanda è stato immediatamente smentito dal collega di opposizione Rutelli, il quale, in un intervento non meno accorato, ha espresso la convinzione che il provvedimento in discussione non sarebbe mai diventato legge, ricordando a tutti noi l'esistenza di un secondo passaggio parlamentare prima del vaglio del Capo dello Stato di un eventuale giudizio di costituzionalità: altro che regime. Vede, senatrice Bassoli, parlando del regime di Sesto San Giovanni il collega Gasparri ha voluto innanzi tutto evidenziare che esistono zone d'Italia, ed è un fatto, nelle quali la maggioranza nel dopoguerra non è mai cambiata, e quella alternanza fisiologica che è la regola aurea della democrazia è ancora sconosciuta. Di «sistema Sesto», d'altra parte, parla oggi anche il «Corriere della Sera», che titola proprio così! Il Capogruppo del PdL ha voluto evidenziare anche come non sia un caso se in queste situazioni iniziano ad emergere possibilità di malgoverno e dubbi sull'onestà di alcuni amministratori che in tali contesti hanno operato. Perché proprio Sesto San Giovanni? Perché dal 1946 al 1962 è stato sindaco Oldrini,

prima PCI e poi Partito Democratico della Sinistra; dal 1994 al 2002 Penati, prima Alleanza dei progressisti e poi L'Ulivo; dal 2002 ad oggi Oldrini, prima Democratici di Sinistra e poi Partito Democratico. Questo non significa, naturalmente, che tutti gli amministratori della storia di Sesto San Giovanni siano stati cattivi amministratori. Ve ne saranno stati anche di ottimi, ma sfido chiunque a sostenere che in quella città vi sia mai stato quel ricambio d'aria utile a prevenire e impedire le incrostazioni del potere. Noi siamo garantisti con tutti, e lo abbiamo dimostrato proprio in quest'Aula. Non siamo però disposti ad essere oggetto di accuse unilaterali fondate su un complesso di superiorità che non ha ragione di essere. La lettera che il segretario del suo partito ha inviato in tal proposito al «Corriere della Sera», collega Bassoli, è un'interessante cartina di tornasole. Bersani, bontà sua, ha affermato che la presunta diversità del PD non è una diversità antropologica. ha, cioè, con tutto il rispetto, scoperto l'acqua calda, perché se si giungesse a negare il principio per cui non esistono diversità antropologiche, si arriverebbe al razzismo fino ai campi di sterminio. Bersani, quindi, si è rifugiato in una proclamazione di diversità politica che, in effetti, forse esiste. Ed è la seguente. Se è vero che la natura umana è una, che ci sono uomini buoni e cattivi, e spesso buoni e cattivi insieme, è certamente possibile, e anzi quasi normale, che possano esserci casi personali e individuali di corruzione nelle file di ogni partito, anche nel mio partito, e laddove la magistratura li scopra, la giustizia deve andare fino in fondo. Rispetto a questa situazione il PD è in effetti diverso. La diversità del suo partito, senatrice Bassoli, da quanto sta emergendo, risiede forse nel fatto che la corruzione potrebbe avere carattere strutturale, legato cioè a quella mancanza di ricambio, a quella stratificazione, a quel consolidamento dei meccanismi di potere che presentano, appunto, connotati di regime. Senatrice, è questo che il presidente Gasparri ha evidenziato con il suo intervento. Forse su questi temi varrebbe veramente aprire tra noi un confronto. È altrettanto evidente che nessuno ha mai inteso offendere la città di Sesto San Giovanni, tanto meno i suoi abitanti. Tutt'altro. Non vorremmo nemmeno ricordare cosa hanno dovuto ascoltare le mura della Camera in questa legislatura, quando il Capo del Governo e *leader* della maggioranza è stato gentilmente definito: «Stupratore della democrazia», «Serpente a sonagli». «Non uno dei tanti tentacoli della piovra, ma la testa della piovra», retta da una «maggioranza farlocca, farlocca, venduta, comprata o ricattata». E non vado oltre. Nella concitazione di una discussione parlamentare quel riferimento a Sesto San Giovanni ha significato semplicemente che noi non ci facciamo dare lezioni e che non abbiamo complessi di inferiorità. Dopo anni di egemonia culturale della sinistra, anche questa è una conquista che rafforza la democrazia e allontana i rischi di regime.

Faccio un intervento di metodo, perché capisco l'intervento della senatrice Bassoli, capisco un po' meno, non nei contenuti, l'intervento del collega collega Quagliariello, che evidentemente sapeva perfettamente su che cosa doveva intervenire e ha potuto spiegare il suo punto di vista. Presidente, lei deve dare garanzie a tutti di intervenire e di potersi preparare

su parere conforme di tutti i Capigruppo, la Presidenza all'inizio della legislatura ha deciso di far svolgere questi interventi a fine seduta. In via del tutto eccezionale, su richiesta espressa della senatrice Bassoli, che mi ha inoltrato una lettera formale, la Presidenza ha voluto derogare a questa intesa in relazione in relazione anche all'intensità dei contenuti e del clima che si era determinato, avendo avuto anche modo di apprendere notizie in ordine a querele, denunzie che sarebbero state inoltrate nei confronti del dichiarante. Proprio perché ci si è resi conto della straordinarietà dell'evento, e proprio per dare la sensazione in Aula subito che nessuno dei componenti di quest'Assemblea credo avesse potuto minimamente immaginare di offendere la storia, i cittadini e le istituzioni di questo paese,

Se non ha ritenuto opportuno informare tutti gli altri Capigruppo, la Presidenza l'ha fatto soltanto in perfetta buona fede, senza minimamente voler mancare di rispetto al dovere di informazione degli altri Gruppi, ritenendo che si trattasse di una vicenda che toccava le dichiarazioni di due esponenti di Gruppi diversi, e non invece un tema politico che meritasse il coinvolgimento di tutte le forze politiche, così come spesso avviene e come voi potete verificare, tanto che intervenite in ogni momento in cui ce n'è la necessità. **Sui

Ho convocato la Conferenza dei Capigruppo per domani alle ore 12 - in maniera che avremo acquisito la tempistica che si sarà data la Camera con la Conferenza dei Capigruppo delle ore

Signor Presidente, ribadisco in Aula la relazione scritta, riservandomi semmai alcune considerazioni all'esito del dibattito che si terrà successivamente. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, già da alcuni anni il Senato della Repubblica ha intrapreso una politica di rigorosa gestione del proprio bilancio interno, resa necessaria sia dal dovere, per le più alte istituzioni repubblicane, di rappresentare verso la collettività un esempio nel corretto utilizzo del denaro pubblico, sia dal contributo che anche il Senato deve offrire al complesso percorso di risanamento dei conti pubblici, funzionale al rispetto degli impegni presi nell'ambito delle procedure del Semestre europeo che impone al nostro Paese il raggiungimento del pareggio di bilancio entro il 2014. Il cammino del risanamento, reso difficile dalla congiuntura economica europea e mondiale, ha trovato uno dei principali passaggi nell'approvazione della recente manovra di stabilizzazione finanziaria contenuta nel decreto-legge n. 98 del 2011. In questo contesto, risulta pertanto condivisibile la scelta dei senatori Questori di modificare il progetto di bilancio, precedentemente approvato dal Consiglio di Presidenza lo scorso 7 giugno, per recepire da subito alcune delle misure di riduzione della spesa contenute nel decreto-legge n. 98 del 2011, che si aggiungono a quelle già adottate in conseguenza della manovra effettuata con il decreto-legge n. 78 del 2010. Rinviando alla relazione di accompagnamento dei documenti di bilancio per un esame più dettagliato dei dati, appare utile ricordare come i risultati di consuntivo contenuti nel rendiconto delle entrate e delle spese per l'anno finanziario 2010 evidenzino un andamento positivo della gestione, con riferimento agli obiettivi di contenimento della spesa del Senato: infatti, la spesa complessiva, rispetto al dato consuntivo dell'esercizio 2009, è stata inferiore al tasso di inflazione programmato. Quest'azione di contenimento dei dati di bilancio si accentuerà nel prossimo triennio attraverso una serie di interventi, già predisposti dal vertice politico dell'Amministrazione, finalizzati a mantenere invariato, per i prossimi tre anni, il costo complessivo dell'Istituzione a carico del bilancio dello Stato e, anzi, consentendo un contributo positivo del Senato a favore del bilancio statale di 120 milioni di euro nel prossimo triennio. L'ampia relazione di accompagnamento al bilancio preventivo per l'anno 2011, contenente la puntuale illustrazione delle singole misure intraprese per il raggiungimento del risultato sopra ricordato, mi consente di non soffermarmi sul merito di tali interventi e dare invece conto di alcune delle questioni sollevate nella riunione dei Presidenti delle Commissioni permanenti. In primo luogo è stata sottolineata la necessità di elaborare documenti contabili che rendano ancor più trasparenti e facilmente leggibili i dati di bilancio, anche al fine di mettere in condizione la pubblica opinione di comprendere la politica di rigore intrapresa in questi anni; è stata altresì sottolineata l'esigenza di predisporre un bilancio di funzionamento, che renda più chiaro il confine tra le spese obbligatorie e quelle di funzionamento in senso proprio. Inoltre, nel riconoscere il contributo responsabile e significativo fornito dal personale all'azione di risanamento, si è posto l'accento sulla necessità di proseguire nella graduale riduzione del numero dei dipendenti che, già sceso dal 2006 ad oggi, dovrebbe diminuire di un ulteriore 25 per cento nei prossimi sette anni. Deve poi proseguire un'azione di razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa, sia ai fini di una migliore allocazione delle risorse umane sia allo scopo di evitare duplicazioni di servizi tra i due rami del Parlamento, con particolare riferimento all'attività di studio e documentazione, nell'intento, tuttavia, di preservare la qualità delle prestazioni offerte. Si è posto poi l'accento sulla necessità di proseguire sulla strada intrapresa del più deciso passaggio al supporto informatico dell'attività svolta attualmente attraverso i documenti cartacei. In conclusione, come ribadito dal Collegio dei senatori Questori, il progetto di bilancio 2011 rappresenta un ulteriore passo in avanti nella gestione rigorosa delle risorse e rende visibile il tentativo di conciliare l'obiettivo prioritario del contenimento della spesa con la piena funzionalità con la piena funzionalità dell'attività parlamentare dell'istituzione democratica.

pochi giorni or sono, il Consiglio di Presidenza ha approvato definitivamente il progetto di bilancio per l'esercizio 2011, apportando al testo originario una serie di modifiche, per alcuni aspetti anche consistenti, in conseguenza di quanto previsto dal recente decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in materia di stabilizzazione finanziaria. Il provvedimento in questione, adottato in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e delle esigenze di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, reca una serie di disposizioni (sull'indennità parlamentare, sulla disponibilità di taluni *benefit*, sulla devoluzione di risparmi conseguiti dagli organi costituzionali, sulla normativa in materia di rimborso ai partiti delle spese elettorali, sull'istituzione di un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici) destinate tutte ad avere ricadute dirette o indirette sul nostro bilancio e che vanno ad aggiungersi alle misure che furono adottate in conseguenza delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010, delle quali si dà ampiamente conto nella relazione di accompagnamento ai documenti di bilancio in esame. Alla luce delle norme sopra richiamate, i senatori Questori, d'intesa con il Presidente del Senato, e dopo essersi incontrati e confrontati con i colleghi deputati Questori, hanno valutato l'esigenza di proporre l'immediata adozione di talune misure di adeguamento della normativa interna ovvero di recepimento sostanziale delle norme sopra descritte: una parte delle misure riguarda i senatori e gli ex parlamentari, l'altra concerne il personale in servizio e in quiescenza. Proprio questa ultima parte ha reso necessaria l'attivazione da parte della Rappresentanza permanente delle procedure prescritte dagli articoli 100 e 101 del Testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione per il personale. Tali nuove misure (la cui quantificazione ammonta complessivamente a quasi 61,3 milioni di euro) consistono: nella riduzione della dotazione ordinaria; nella mancata applicazione alle retribuzioni del personale dell'incremento del 3,2 per cento corrisposto invece ai dipendenti della Camera; nel recepimento del contributo di perequazione del 5 e del 10 per cento sulle pensioni più elevate degli ex dipendenti e nell'applicazione dello stesso contributo ai vitalizi più elevati degli ex senatori; infine, in ulteriori riduzioni degli oneri locativi. Il pacchetto di misure appena descritto si dovrà completare con ulteriori mirati interventi che i senatori Questori intendono proporre al Consiglio di Presidenza prossimamente, al fine di dare autonoma e corretta attuazione sia ad altri indirizzi di contenimento della spesa previsti nella manovra appena approvata dal Parlamento (in funzione, tra l'altro, di un riordino della disciplina della indennità parlamentare e delle competenze accessorie) sia al processo di riorganizzazione e razionalizzazione della struttura amministrativa. Non v'è dubbio, tuttavia, che il principale intervento che nell'immediato si ritiene di adottare riguarda il versante delle entrate, riducendo, analogamente alla Camera dei deputati, la richiesta di dotazione finanziaria per gli anni 2012 e 2013 allo stesso valore del 2011, in modo da mantenere per ulteriori 2 anni il *trend* di "crescita zero" già avviato con l'esercizio finanziario in corso. Tale misura - che da sola consente un risparmio per il bilancio dello Stato di ulteriori 24 milioni di euro circa, dei quali 7,9 milioni rispetto a quanto previsto inizialmente per il 2012 ed ulteriori 15,9 milioni rispetto al 2013 rappresenta un vincolo particolarmente gravoso (cui si farà fronte rimodulando nel tempo l'avanzo di gestione accertato con l'approvazione del rendiconto di esercizio 2010), considerato che le provviste finanziarie del nostro bilancio sono costituite essenzialmente dalla dotazione ordinaria (88 per cento), laddove, sul versante delle uscite, gran parte della spesa ha carattere obbligatorio: il recepimento di un vincolo così stringente impone di rafforzare l'impegno a perseguire l'obiettivo di contenimento e razionalizzazione della spesa. L'altra misura di particolare rilievo che il Senato si impegna ad applicare consiste nel cosiddetto contributo di perequazione del 5 e del 10 per cento sia sui vitalizi degli ex parlamentari, che sulle sulle pensioni degli ex dipendenti che superano, rispettivamente, i 90.000 ed i 150.000 euro: tale contributo recherà un gettito di circa 1,1 milioni di euro 2,9 milioni di euro nel 2013 e 3,2 milioni di euro nel 2014, che verrà integralmente versato all'erario. Senza entrare in questioni relative alla natura dei vitalizi e nelle more di una riforma complessiva dell'istituto, sotto il profilo politico generale appare opportuno che anche i parlamentari cessati dal mandato (così come i dipendenti in quiescenza) contribuiscano al generale impegno per il contenimento della spesa pubblica, cui già danno il loro apporto i parlamentari in carica e i dipendenti delle Camere. Considerando anche gli interventi adottati alla fine dell'anno 2010 2010 (riduzione delle retribuzioni più elevate del personale, riduzione delle competenze accessorie dei senatori, mancato adeguamento contrattuale di retribuzioni e pensioni, risparmi per dematerializzazioni degli atti parlamentari e per dismissione di locazioni) ed un arco temporale comprensivo dell'anno 2014, l'effetto congiunto dell'intera manovra adottata dal Senato, tra la seconda metà del 2010 ed oggi, ammonta ammonta complessivamente a 120 milioni di euro, tra riduzioni di spesa e diminuzioni di trasferimenti statali, avuto appunto riguardo anche alle misure già decise lo scorso anno per 58,7 milioni di euro. A differenza di qualche ingiusta valutazione critica emersa in qualche ordine del giorno, bisogna invece sottolineare che il risultato di riduzione del bilancio dello 0,34 per cento rispetto allo scorso anno che si raggiunge nel 2011 è di singolare, direi storica, portata: è la prima volta, infatti, che nella dinamica delle spese finalmente si scende sul serio. Certo, è appena l'inizio, ma non è neanche poi così poco se si considera un tasso di inflazione reale intorno al 2,7 per cento annuo. È il segno di un cambiamento di tendenza, di rotta, che non c'è mai stato prima e che si rafforzerà grazie proprio alle misure di cui la Presidenza e i senatori Questori hanno inteso proporre l'adozione. Considerando che se ne fa anche oggetto di un sondaggio televisivo, consentitemi di spendere, infine, qualche parola, in particolare, riguardo a ciò che è stato fatto nel corso degli ultimi anni in materia di ridimensionamento del trattamento complessivo dei senatori, al fine di partecipare al generale sforzo di riduzione della spesa pubblica. Segnalo solo le più importanti novità. Con la legge finanziaria 2006, l'importo dell'indennità parlamentare è stato ridotto strutturalmente del 10 successivamente, la legge finanziaria 2008 ha bloccato per cinque anni gli incrementi dell'indennità spettanti a diritto vigente, dal 2008 al 2012. Per effetto di queste decisioni, attualmente l'importo lordo dell'indennità dei senatori è di poco superiore ai 12.000 euro mensili, cioè al 70,59 per cento del trattamento complessivo massimo dei magistrati di riferimento, all'ultimo aumento biennale, pari ad oggi a euro 14.756 euro mensili. Con la deliberazione del Consiglio di Presidenza, poi, dal 1° gennaio 2011 i rimborsi spesa forfettari sono stati ridotti complessivamente di 1.000 euro al mese (500 euro decurtati dalla diaria di soggiorno e 500 dal contributo per il supporto dell'attività dei senatori). Nel 2007 è stata approvata una riforma degli assegni vitalizi, che ha sensibilmente ridotto la misura di tali prestazioni e ha raddoppiato il periodo minimo di mandato richiesto per maturare il diritto all'assegno vitalizio: fino alla XV legislatura erano sufficienti 2 anni e 6 mesi - con il pagamento dei contributi figurativi per il completamento del quinquennio contributivo - mentre dalla legislatura in corso sono richiesti almeno 5 anni effettivi di mandato, in una o più legislature. Già nel 1997 era stato elevato il requisito di età per fruire del vitalizio, che in precedenza variava da un minimo di 50 a un massimo di 60 anni, a seconda del numero di legislature svolte, mentre ora l'intervallo è tra i 60 e i 65 anni. a partire dal 1° gennaio 2010, sono state notevolmente ridotte le facilitazioni di viaggio a favore degli ex senatori, con la soppressione di ogni rimborso dei pedaggi autostradali e con l'introduzione di un tetto annuale per i viaggi aerei e ferroviari sul territorio nazionale. Tali benefìci sono stati altresì limitati a un periodo di 10 anni dalla cessazione dal mandato, oltre il quale cessa ogni facilitazione. Concludo ribadendo la fermezza con la quale la Presidenza e i senatori Questori intendono proseguire nella rigorosa gestione delle risorse di bilancio, attenti all'obiettivo prioritario del contenimento della spesa e determinati a portare a compimento e ad integrare gli interventi necessari per assicurare la piena funzionalità, efficienza ed economicità dell'attività parlamentare. *(Applausi

*(PD)*. Signor Presidente, per usare parole semplici, ritengo che il bilancio sia del tutto inadeguato alle aspettative dell'opinione pubblica e alle necessità inerenti allo stato della finanza pubblica.

Penso che sia stato un grave errore non aver inserito nella manovra, come noi avevamo proposto, delle misure più rigorose sui costi della politica, per una questione di equità, ma anche di autorevolezza, per affrontare le tante altre sacche di privilegio che ci sono nella società italiana. Ricordo per memoria, ad esempio, che il sistema camerale italiano prevede la partecipazione in oltre 1.800 società, ognuna con il suo consiglio di amministrazione; e ricordo - sempre per memoria - che recentemente due soli banchieri hanno ricevuto tra buonuscite, liquidazioni e altro, la cifra di 60 milioni di euro, cioè più del costo dell'intero Senato. Sappiamo che dietro la questione dei costi si nasconde una questione molto più ampia: una politica che viene avvertita come lenta e lontana e una rappresentanza indebolita dall'ignobile legge elettorale che avete imposto al Paese. Penso che con il bilancio si possa cogliere l'occasione di ridare reputazione alla funzione parlamentare e maggiore efficienza alla macchina del Senato. Mi consentirà, signor Presidente, di rivolgere a lei una critica, che naturalmente potrà spartire con il presidente Fini.

che noi godiamo di un trattamento sanitario talmente favorevole da costare alla comunità oltre 10 milioni di euro. Noi sappiamo che questa notizia è palesemente falsa, perché il sostegno sanitario è completamente alimentato dai versamenti obbligatori dei parlamentari. Da parte vostra c'è stato solo silenzio: mai un intervento di correzione a difesa della onorabilità dei parlamentari, non ricordando neppure le cose fatte, che ha ricordato da ultimo il senatore Franco. Si tratta di ricostruire un rapporto con l'opinione pubblica, mantenendo ciò che va mantenuto. Va benissimo l'equiparazione a livello europeo, ma bisogna difendere nell'opinione pubblica con argomentazioni e non con silenzi corrucciati. Occorre cambiare ciò che va cambiato. Diaria e contributo di supporto devono essere legati alle presenze reali in Aula e in Commissione

fino a che punto è condivisibile che in Aula ci si occupi talvolta di mozioni che - come dire? - lasciano il tempo che trovano e che le Commissioni, dove potremmo approfondire gli argomenti,

quanto uso si fa degli aerei di Stato da parte di parlamentari. Io sono qui dal 1996 e non so come sia fatto un aereo di Stato. Spero di non essere l'unico. Dobbiamo cambiare il vitalizio. Così com'è, esso è espressione di un altro tipo di società. Certo, giuridicamente non è una pensione, ha un'altra natura, ma deve avere un meccanismo uguale a quello previsto per tutti gli altri cittadini italiani.

possibilmente un *self-service* - in cui sia possibile consumare un pasto rapido; e non deve essere a carico dei cittadini, ma interamente a carico dei senatori e dei dipendenti del Senato, che in larga parte se lo possono permettere. Il secondo punto attiene al recupero di efficienza. Signor Presidente, la seconda istituzione dello Stato - chiamiamo così il nostro Senato - approva il bilancio preventivo

Penso di no. I colleghi che mi seguiranno credo faranno molte proposte. Io mi soffermo su tre punti. In primo luogo, la spesa per il personale addetto alle segreterie particolari cresce da 13,5 a 14,9 milioni,

Dove va a finire la terzietà della pubblica amministrazione, che è un grande valore del Senato e della Camera? C'è ovviamente una mancata trasparenza e anche - consentitemi - l'alimentazione della precarietà di un ceto che resta legato alle contingenze della politica, e quando cambiano i senatori Questori, quando cambiano i Presidenti, c'è il problema della ricollocazione. Quindi, si alimenta un ceto politico, c'è una maggiore richiesta di logistica, di attrezzature, e si realizza anche una inaccettabile disparità tra di noi: un numero ristretto di senatori gode di servizi profondamente diversi da quelli di tutti gli altri senatori. senatori. Dal bilancio di quest'anno risulta che i risparmi dati dalle riduzioni delle nostre competenze vanno interamente ad alimentare l'aumento della disponibilità di risorse da parte delle segreterie particolari. Questo certamente non va bene. C'è il capitolo del contributo dei Gruppi: benissimo, è una condizione di libertà, però insindacabilità non può vuol opacità. I soldi pubblici restano tali anche quando entrano nelle casse dei Gruppi. Per questo ho presentato un ordine del giorno che prevede la presentazione di un bilancio tipo e una rendicontazione. voci: comunicazione istituzionale, cerimoniale, rappresentanza. Si può fare molto di più. I Comuni non hanno più spese di comunicazione e di rappresentanza. Per quale motivo noi dobbiamo conservarne un livello così elevato? Si può fare molto di più. Si parla di antipolitica, ma guardate che l'antipolitica talvolta è nostalgia per la buona politica. Concludo con un messaggio. Don Primo Mazzolari, nel 1948, scrisse una lettera ai parlamentari neoeletti dicendo: «Non potete fare molto perché non vi fu data, con il suffragio, l'onnipotenza. Sarà bene però che tutti vedano che tutto ciò che si poteva fare l'avete fatto con estrema buona volontà; dovete dar vita a un nuovo costume politico». È un messaggio di grande attualità: dobbiamo dar vita a un nuovo costume politico. Questo bilancio è troppo timido rispetto a tale impegno. Signora Presidente, colleghi, a me dispiace che il Presidente sia andato via, ma annunciare che non si voterà questa sera mi sembra quasi abbattere l'interesse intorno a questo dibattito, credo volutamente. Mi dispiace dirlo, ma è così. Penso che siamo oggi in un momento in cui il sano trasversalismo tra le forze politiche deve avere la meglio su una lottizzazione stupida e ridicola che da qualche anno si porta avanti nella gestione del bilancio del Senato.

io non mi sento tale, non mi sento un parassita, mi sento un parlamentare che ha inteso lavorare, ha inteso partecipare al dibattito, e credo che questi parlamentari, che sono quasi tutti, andavano difesi dalla nostra dirigenza.

con una conferenza stampa, con una trasparenza, con un ufficio apposito, dicendo, senza paura, come si doveva, qual è la verità e qual è la bugia, perché nessuno si vergogna di prendere 12.000 euro al mese, nessuno si vergogna di determinate cose, ma ci vergogniamo certamente di determinati *benefit*, che possono essere assolutamente cancellati. Ecco perché oggi bisogna fare l'operazione di verità:

Io non ho potuto prendere atto dei nomi dei collaboratori, per esempio, dei nostri Vice Presidenti e dei nostri Segretari. Credo che tenerli nascosti sia una cosa che non va.

recuperare capacità e credibilità presso la nostra gente. Al di là del tecnicismo, signori Questori del bilancio, sono vere le cose dette dal relatore, ma non noto nessun respiro programmatorio; cioè non noto in questo bilancio nessun afflato

mi dispiace dirlo - alcuni risparmi sono dovuti alla manovra finanziaria e non sono un merito di questa Amministrazione. oggi viviamo una crisi tremenda, non lo dobbiamo fare perché dobbiamo adeguarci ai sacrifici di tanta gente, ma perché va fatto un risparmio

che avete approvato in questi giorni vanno a danno soprattutto dei meno abbienti, di chi ha un reddito inferiore.

Attraverso gli anni tutte le forze politiche ci hanno messo qualche mattone. Oggi tutti insieme dobbiamo cercare di invertire la rotta, e non con l'acquiescenza a determinati benefici che si hanno. Per esempio, esempio, avete mai pensato che era opportuno che oggi si annunciasse che vanno modificati i Regolamenti? Non si parla di trattamenti economici e di dimezzamento dei trattamenti economici, per esempio, dei Segretari,

la casta nella casta. Si sta creando questo: noi, come senatori, siamo tutti uguali: ognuno ha un ruolo diverso dall'altro, ma non si possono favorire privilegi. Ecco perché bisogna fare delle riforme regolamentari. Vi sembra giusto che questo Senato abbia quattro Vice Presidenti

nell'intento di non danneggiare il dipendente e, al tempo stesso, di non favorire nessuna piccola casta che utilizza e mortifica anche il personale. Il personale a suo tempo deliberato nel 1993 deve lavorare, e deve farlo con dignità:

sono un po' meravigliato che le spese di rappresentanza e per il cerimoniale ammontino a 2 milioni e 200.000 euro: mi sembrano eccessive. Così come l'abbonamento alle agenzie. Ha ragione il relatore: bisogna assolutamente mettersi d'accordo con la Camera dei deputati,

nazionale. Credo che sia una richiesta di tutti i senatori che lavorano: non è possibile non legare una parte dell'indennità

perché al Parlamento guardano anche le Regioni, che spesso lo scimmiottano. Per esempio, nella mia Regione vi sono 14 Gruppi; in Basilicata, 13 Gruppi con 30-40 consiglieri. Credo che ciò sia assurdo, perché si legano al Parlamento! Diamo quindi anche cattivi esempi. Credo che facendo questo, andiamo a fare anche un'opera di recupero di credibilità della politica, che dobbiamo assolutamente portare avanti per poter riprendere il ruolo prestigioso del Parlamento italiano.

Il primo punto che voglio sottolineare è che dovremmo essere in grado - e molto spesso non lo siamo - di fare una differenza tra i costi della politica e i costi della partitocrazia: cari colleghi, sono due cose diverse! avere il coraggio di rivendicare che la nobiltà della politica costa e ha bisogno di essere sostenuta, ma discutendo come accettando che certamente molte delle degenerazioni partitocratiche hanno finito oggi per mangiare buona parte di questa credibilità. Non voglio sembrare quella che parla d'altro, e neanche voglio far parte di schiere, che pure vedo particolarmente appassionate in questi giorni: mi auguro che la loro passione possa essere più continuativa nel tempo e meno sporadica. Non amo rincorrere né Facebook né Twitter; non amo tanto meno rincorrere o usare la demagogia. Ho l'orgoglio di aver proposto da tanto tempo, come radicale, un metodo - e uno solo - per affrontare questo problema: quello della trasparenza, a cominciare dall'anagrafe pubblica degli eletti.

che lo stato patrimoniale possa essere reso pubblico da ciascuno di noi tramite Internet, ma voglio informare tutti quanti che sono solo 50 i senatori che hanno mandato la liberatoria e che solo 17 hanno concluso le procedure. Quindi, va tutto bene - per carità! - quello che sento dire in questi giorni, ma andrebbe altrettanto bene, e forse meglio, se cominciassimo da noi, tanto per gradire. Si tratta di una possibilità e di una responsabilità che questa amministrazione ha messo a disposizione di tutti. Constato, però, che solamente 17 ne hanno voluto in qualche modo usufruire. Qualcosa non mi torna, allora, in tutta una serie di furori attuali.

luogo, esistono ancora buchi di non trasparenza che devono essere chiariti, a cominciare - per esempio - dal contributo per le attività di collegio. I Questori sanno, in quanto l'ho detto fino allo sfinimento in Consiglio di Presidenza,

amministrarla nel modo più oculato, così come dobbiamo fare con tutto il denaro pubblico. Bisogna però sapere di cosa stiamo parlando, poiché l'approccio di molti mezzi di informazione ai cosiddetti costi della politica non ci aiuta, quanto diffonde costantemente dei veri e propri falsi accompagnati da mistificazioni e distorsioni che sfociano in una indignazione irta di insulti, la quale non può che essere in mala fede quando viene da chi fabbrica e propaga tali falsità. Orbene, di questi quasi 527 milioni, sottratti i risparmi che verranno versati allo Stato e le somme che rientrano nelle casse pubbliche immediatamente sotto forma di imposte sul reddito, il vero costo di questa istituzione per i contribuenti è di 400 milioni, pur includendo parecchi milioni di IVA che il Senato paga. Si tratta dello 0,05 per cento della spesa pubblica, 56 centesimi al mese per ogni contribuente. Insomma, l'intero Senato costa a un singolo cittadino molto meno di un decimo, forse un ventesimo dell'iscrizione al sindacato. Con il costo di una copia del libro «La Casta» un cittadino si campa l'intero Senato per quasi tre anni. Ma di questi 400 milioni solo 114 sono destinati ai senatori, inclusi i rimborsi, i vitalizi per gli ex, le spese di trasporto e di ristorazione: fa 16 centesimi al mese per italiano, lo 0,014 per cento della spesa pubblica,

A ogni italiano, il singolo senatore costa un centesimo ogni 20 mesi. È perciò degna di nota l'abilità di chi, facendo sensazionalismo su queste cifre, di solito truccate, riesce a guadagnare qualche milione di euro. Detto questo, è nostro preciso dovere agire con la diligenza del buon padre di famiglia, come dice il codice civile, e, vorrei aggiungere, della buona madre di famiglia, per contenere le spese, per quanto siano una piccolissima frazione del bilancio dello Stato. Ecco perché le nostre indennità sono bloccate dal 2008, dopo che nel 2006 erano state ridotte del 10 per cento. La diaria e il contributo di supporto sono rimasti bloccati dal 2001 per poi essere decurtati di mille euro al mese proprio all'inizio di quest'anno. Nel complesso, il valore reale dell'indennità netta è sceso del 24 per cento rispetto al 1994. La diaria e il contributo di supporto sono scesi del 28 per cento in dieci anni. Vale anche la pena di ricordare che la legge del 1965, che regola, sulla base della Costituzione, le nostre indennità, ci equiparava al presidente di sezione della Corte di cassazione. Nella realtà, oggi quel presidente prende oltre il 41 per cento più di noi, con il vantaggio peraltro di non ricevere insulti dalle prime pagine dei giornali. La stessa legge del 1965 prevedeva che gran parte dell'indennità fosse esente dalle imposte sul reddito, ma la legge finanziaria del primo Governo Berlusconi cancellò completamente ogni esenzione. È curioso notare che negli anni in cui veniva creato l'immenso debito pubblico che affligge noi e le generazioni che ci seguono, i parlamentari avevano un trattamento economico assai più pingue, ma la stampa non si indignava: forse aveva le sue buone ragioni. Dunque, il nostro costo è la duemillesima parte della spesa pubblica, e i nostri compensi sono scesi di un quarto negli ultimi 10-20 anni. Ma tanti ben pagati giornalisti, e a volte anche i loro benissimo pagati direttori continuano a ripetere che noi guadagniamo molto più dei nostri colleghi del resto d'Europa. Se così fosse, conterebbe poco che i nostri compensi siano scesi. Il fatto è che quegli stessi giornali che ci additano come i Paperoni d'Europa, quando il mese scorso abbiamo votato, nell'ambito della manovra finanziaria, l'adeguamento del nostro trattamento ai sei principali Paesi dell'area euro, ci hanno accusato di non aver fatto alcun taglio. È evidente che o mentono nel dire che guadagniamo più degli altri o mentono nel dire che adeguandoci agli altri non ci riduciamo i compensi. In realtà, mentivano in entrambi i casi, perché non è vero, come vedremo, che abbiamo un trattamento economico più alto degli altri grandi Paesi. E non è neppure vero che non subiremo alcuna riduzione, visto che tra i sei principali Paesi dell'area euro, ce ne sono quattro con popolazione e prodotto interno lordo inferiori all'Italia, anche di cinque o sei volte, ed è normale che i parlamentari abbiano trattamenti economici più bassi. Ma molti giornalisti di valore - di valore nel senso che sono molto pagati *(Applausi dal Gruppo PdL)*- scrivono un giorno sì e l'altro pure che siamo i più pagati d'Europa, molto più pagati degli altri. Un messaggio semplice, che colpisce l'opinione pubblica. Guardiamo allora al caso più vicino a casa nostra: la Francia. Stessa popolazione, 32 parlamentari in meno, ma tra questi i senatori sono 343, 28 più di noi. Vale la pena ricordare che i senatori francesi non sono votati dal popolo, ma dagli eletti del loro collegio. Dunque, niente costi di campagna elettorale. La loro indennità netta è circa 300 euro superiore a quella nostra. Se poi superano i 15 anni di mandato, fanno un balzo in avanti di 1.218 euro, perché non più soggetti a una certa ritenuta. A differenza di quanto accade in Italia, possono poi cumulare indennità derivanti da altre cariche pubbliche, sia pure con il limite di 2.757 euro al mese. In Francia moltissimi parlamentari, infatti, sono anche sindaci, anche perché, con la nostra stessa popolazione, hanno 36.000 Comuni contro i nostri 8.000. Si dirà allora che c'è il trucco: i senatori italiani avranno trattamenti accessori maggiori. Vediamo: i nostri colleghi francesi hanno 6.412 euro netti al mese per spese di mandato; noi, sommando la diaria ed il contributo di supporto, li superiamo di 1.268 euro. Ma al posto di quei 1.268 euro i senatori transalpini hanno 7.548 euro per il personale alle loro dipendenze; in più, gli oneri del datore di lavoro restano a carico del Senato, cosa che noi non abbiamo, un vantaggio calcolabile in almeno 4.000 euro. Per quanto riguarda le altre spese, il trattamento è equivalente. In più i membri del Senato francese si vedono rimborsare le spese d'albergo a Parigi nei giorni di seduta e godono di prestiti a tasso agevolato al 2 per cento, cose del tutto sconosciute Si dirà, chissà quanto lavorano a Parigi! Glielo chiederemo al più presto; però ci vuole un po' di pazienza, perché la scorsa sessione si è chiusa il 13 luglio e la prossima inizierà l'11 ottobre! Tutte queste cose si possono molto facilmente trovare nel sito Internet del Senato francese, cosa probabilmente troppo faticosa per i nostri principi dell'informazione sensazionalistica. i documenti che attestano questi ed altri dati, perché gli atti del Senato riportino la verità *per tabulas*. Visto che si cita così spesso l'estero, vorrei ricordare che in altri Paesi, i giornalisti che diffondono scientemente (ma anche non scientemente) notizie false, specie sulle istituzioni, di solito perdono il posto, generalmente dimettendosi loro stessi per evitare l'umiliazione del licenziamento. Insomma, i senatori francesi, per sé e per il loro personale, hanno a disposizione circa 10.000 euro al mese più di quelli italiani, ma ci viene detto che noi siamo i più i pagati. Vogliamo parlare dei deputati tedeschi? Basti dire che solo di diaria prendono 1.000 euro al mese più di noi e che per il personale hanno a disposizione 14.712 euro al mese, tre volte e mezzo il nostro contributo di supporto; hanno tutti l'auto pubblica a disposizione per servizio in Berlino, mentre da noi ce l'hanno solo una ventina di senatori e deputati con particolari cariche; hanno hanno il vitalizio, cui hanno diritto anche dopo un solo anno di legislatura, senza pagare i contributi pensionistici. Ecco perché, come anche i francesi, hanno un'indennità lorda più bassa della nostra, ma un netto superiore. Un ennesimo gioiello del giornalismo d'autore è stata l'affermazione secondo la quale Senato e Camera italiani costerebbero 100 milioni più dei loro corrispondenti di Washington. Chi ha letto questa presunta verità assoluta è trasalito: ma come, gli Stati Uniti, più grandi e più ricchi di noi, hanno un Parlamento che costa meno? C'è persino un po' di verosimiglianza, visto che i parlamentari americani sono meno numerosi di noi. Ma anche questa è una balla, forse più spudorata delle altre. Di nuovo, basterebbe controllare su Internet: Senato e Camera degli Stati Uniti costano non 100 milioni in meno, ma 2,3 miliardi in più! Non è strano, dato che i deputati, oltre all'indennità, hanno a disposizione per le loro spese fino a l00.000 euro al mese e i senatori fino a 280.000 euro al mese. Sottolineo "euro" e sottolineo "al E va detto che, a differenza di quanto avviene nei nostri bilanci, il costo del Congresso americano non comprende i vitalizi dei parlamentari e le pensioni dei dipendenti, cosa che vale anche per i principali Parlamenti europei: ecco perché il nostro Parlamento sembra sempre più caro degli altri. Messo in chiaro tutto questo, noi, come Gruppo del Popolo della Libertà, siamo impegnati a continuare sulla strada della riduzione della spesa, come dimostrano le cifre del bilancio approvato in Consiglio di Presidenza che, per il terzo anno consecutivo, non incrementa la spesa in termini nominali e dunque la riduce sensibilmente in termini reali, cosa mai avvenuta prima, neanche per un solo anno, e come dimostra l'ordine del giorno che presentiamo come Popolo delle Libertà con importanti proposte per proseguire la razionalizzazione. Il Partito Democratico, invece, mostra di avere più di una faccia. I suoi autorevoli rappresentanti nel Consiglio di Presidenza hanno approvato con noi un bilancio virtuoso, con importanti misure di risparmio. Del resto, anche noi nella scorsa legislatura approvammo, sotto la Presidenza Marini, dei bilanci contenenti misure di risparmio. Poi, però, i vertici del Gruppo del Partito Democratico presentano un ordine del giorno che sconfessa completamente l'intero Consiglio di Presidenza, inclusi i membri appartenenti al loro stesso Gruppo, disegnando fantasiosi e demagogici scenari. Ora, va bene che questo "PD due" sa che verrà approvato il bilancio approvato anche dal "PD uno" e non questo strampalato ordine del giorno; però un po' di pudore non guasterebbe. Il senatore Morando, uno che conosce i bilanci come pochi e dunque sa molto bene di cosa parla, oggi scrive questo ordine del giorno che attacca frontalmente il terzo bilancio consecutivo in cui si riduce il peso del Senato sui contribuenti. Ma quando toccò a lui essere relatore dell'ultimo bilancio approvato nella scorsa legislatura, il 4 aprile 2007, nella lunga relazione e nella altrettanto lunga replica non pensò di dire una parola sul fatto che le spese del Senato aumentassero del 2,77 per cento, ben oltre il tasso di inflazione. Ieri la spesa saliva ed era tutto a posto; oggi la spesa scende e ci si oppone. Complimenti per la coerenza, ma non crediate di fare fessi gli elettori, che fessi non sono! Il fatto è che i signori della sinistra sui costi della politica sono bravissimi a parlare, ma le cose concrete le abbiamo sempre fatte noi. Siamo noi, che nel primo Governo Berlusconi abbiamo abolito ogni esenzione dalle imposte per l'indennità parlamentare, non voi. Siamo noi che abbiamo ridotto del venti per cento i consiglieri provinciali e comunali in questa legislatura. Siete voi che avete fatto il Governo dei 101 Ministri e Sottosegretari, noi siamo scesi di 40: il 40 per cento Siamo noi che abbiamo approvato dopo un faticoso *iter* parlamentare la riduzione del numero dei parlamentari, che sarebbe già in atto da tre anni se non aveste condotto una feroce campagna contro la modifica della Costituzione, che portò alla bocciatura della riforma con il *referendum* del 25 giugno 2006. Oggi, per Oggi, per nascondere questa evidenza, vi agitate per calendarizzare lo stesso provvedimento. Siamo noi che abbiamo approvato la liberalizzazione dei servizi pubblici locali, per abolire il monopolio e il «magna-magna» delle municipalizzate, con le migliaia di assunzioni clientelari, le nomine dei dirigenti di stampo politico Pensa a Milano! MALAN *(PdL)*. ...sulla gestione degli acquedotti, la raccolta rifiuti e i trasporti locali. Siete voi che con una campagna di menzogne avete convinto gli italiani a bocciare questa riforma, raccontando che avrebbero dovuto pagare per bere alla fontanella pubblica e che l'Italia sarebbe diventata come Cochabamba! Siete voi che nel 1995 lavoraste per bocciare il *referendum* che aboliva il doppio turno alle amministrative, e oggi volete addirittura introdurlo per le elezioni politiche, con un costo di qualche centinaio di milioni per legislatura. E allora, anche oggi, noi ci assumiamo volentieri la responsabilità di fare i risparmi veri, votando un bilancio virtuoso che riduce le spese e votando il nostro ordine del giorno che traccia la strada per ulteriori risparmi ed efficienza per il futuro; e lasciamo volentieri a voi la cinica demagogia, il meschino chiacchiericcio e quell'atteggiamento di cui parla Dante nel XXIII canto dell'Inferno. Signor Presidente, signori Questori, colleghi, nel Paese è in atto una campagna «moralizzatrice» contro la «casta della politica», che ha preso di mira i cosiddetti privilegi dei parlamentari, le indennità ed i vitalizi, non soltanto sulla rete e da parte dei grandi giornali, ma perfino da parte del TGl, il cui direttore Minzolini è sotto inchiesta penale per l'uso disinvolto della carta di credito aziendale. ha dato voce alla rivolta anti-casta, attaccando il bilancio di Camera e Senato quasi fossero la causa principale della voragine del debito pubblico, mettendo alla gogna i parlamentari accusati di «vivere sulle spalle dei lavoratori», quasi ci dovessimo vergognare di essere stati eletti. L'idea che sta avanzando nel Paese è che tutti coloro che ricoprono una carica elettiva fanno parte della casta, che la casta è uno sperpero di denaro pubblico, che deputati e senatori sono troppi, che l'idea di avere due Camere è un lusso: ne basterebbe una con pochi rappresentanti e poi si potrebbe abolire anche quella. Nei tempi in cui emergono collegamenti tra la P4 e la P2, mi torna in mente il Piano di rinascita nazionale di Licio Gelli: svuotare il Parlamento delle sue prerogative di rappresentanza popolare, liquidare il controllo parlamentare sull'Esecutivo, passare ad una Repubblica presidenziale, dare la spallata definitiva alla odiata casta, che rappresenta un intralcio al decisionismo dell'azione politica. I potentati economici e finanziari - proprietari di quotidiani e televisioni con i quali esercitano un potere enorme senza bisogno di confrontarsi con il corpo elettorale i banchieri e le grandi banche di affari, che governano i destini del mondo e che hanno prodotto la crisi sistemica, sono arrivati a ribaltare la realtà dei fatti ha detto anche il senatore Giaretta: 60 milioni di euro per due banchieri, il costo del Senato) e dando la caccia all'untore, ossia Governi e Parlamenti deboli, perché ricattati ed asserviti a disegni superiori. Sparano nel mucchio in un clima culturale pervaso dall'egoismo, da un'etica messa sotto i piedi perché comandata da un utilitarismo economico e dallo strapotere dei *mass media*, con una politica che non è più al servizio degli interessi generali e del bene comune; sparano nel mucchio perché nella notte, come diceva Hegel, tutte le vacche sono nere e tutti i gatti sono bigi. II 28 luglio 1981 Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista Italiano, rilasciò una celebre intervista a Eugenio Scalfari, il direttore de «la Repubblica», in cui sottolineava tematiche che oggi, a 30 anni di distanza, tornano ad essere drammaticamente attuali: l'austerità nei consumi e la questione morale nella politica. "Per noi comunisti la passione non è finita. Ma per gli altri? Non voglio dar giudizi e mettere il piede in casa altrui, ma i fatti ci sono e sono sotto gli occhi di tutti. I partiti sono soprattutto macchine di potere e di clientela: scarsa o mistificata conoscenza, programmi vaghi, sentimenti e passione civile zero. Gestiscono interessi, i più disparati, i più contraddittori, talvolta anche loschi, comunque senza alcun rapporto con le esigenze e i bisogni umani emergenti, oppure distorcendoli senza perseguire il bene comune". Non continuo sull'occupazione, sulla televisione, sui giornali, sul credito bancario. "Molti italiani" - aggiungeva Berlinguer - "si accorgono benissimo del mercimonio che si fa dello Stato, delle sopraffazioni, dei favoritismi, delle discriminazioni. Ma gran parte di loro è sotto ricatto. Hanno ricevuto vantaggi (magari dovuti, ma ottenuti solo attraverso i canali dei partiti e delle loro correnti) e sperano di riceverne, o temono di non riceverne più". le inchieste della magistratura stanno mettendo in luce un sistema di potere e di lotta senza quartiere tra i poteri dello Stato, finalizzato all'esclusivo arricchimento personale. Non si ruba più per il partito; la tangente si è ingegnerizzata: si ruba per se stessi o tutt'al più per le varie cricche che assegnano appalti secretati per impedirne la tracciabilità. La politica è debole e subisce in silenzio i ricatti di oligarchi e tecnocrati, *manager* pubblici, banchieri strapagati, giudici amministrativi spesso ladri di diritti, che possono continuare a esprimere lodi milionari a collaudi ed arbitrati, senza che vi sia conflitto di interessi ed alcun richiamo all'etica pubblica ed alla questione morale, che dovrebbe valere per tutti. Abbiamo presentato alcuni ordini del giorno, alcuni a mia prima firma, riguardanti la gestione dei palazzi, oggetto di perenni lavori di manutenzione, auspicando che possano essere adottati criteri di maggior trasparenza in riferimento all'*iter* delle gare di appalto e della politica immobiliare. Un altro ordine del giorno

poi altre voci di bilancio, come i contratti di locazione, la manutenzione ordinaria dei fabbricati (5.274.000 euro che passeranno a 5.959.000),

oneri non ripartibili (25.785.000 euro). Signori Questori, colleghi, la democrazia e le istituzioni rappresentative hanno un costo funzionale intrinseco

del 50 per cento le spese per l'adozione di sistemi di sicurezza e del 30 per cento degli oneri relativi ai servizi diversi da quelli riferiti strettamente all'attività parlamentare. Signora Presidente, la politica è debole, lo ripeto, perché ricattata da tecnocrati ed oligarchi che si possono permettere di stare in 54 consigli di amministrazione come il presidente dell'INPS - e vengono poi qui a darci lezioni. È sotto gli occhi di tutti una commistione tra politica ed affari, un mercimonio delle nomine pubbliche, un sistema gelatinoso che pervade ogni apparato, soprattutto quando si ricorre alla segretezza degli appalti. Per questa ragione, noi dobbiamo fare di più - abbiamo il dovere di dare risposte ai cittadini in quei capitoli di spesa dove si può e si deve tagliare; ma dobbiamo difendere tutti i costi della democrazia senza distinzione. I diritti non hanno colore politico: ho speso una vita per difenderli, e continuo, e con me molti senatori, a vedere la politica nel senso nobile, ossia al servizio dei cittadini, della collettività e dell'interesse generale. Come tanti altri, non uso l'auto blu non sono mai andato sui "voli blu", ma uso i mezzi pubblici e un motorino, al quale qualche oscuro e frustrato funzionario burocrate voleva impedire l'accesso al Senato,

Quando un funzionario si permette di telefonare ad un senatore per dirgli: «Lei è stato visto con il motorino»... Ma di cosa parliamo? Ma non accetto, signori senatori, di passare per un ladro facente parte di una casta che ruberebbe lo stipendio. Bisogna risparmiare ed asciugare quelle voci di bilancio, rivedere la questione morale

la discussione e il voto sul bilancio del Senato sia un'occasione importante, un'occasione che questa Assemblea può cogliere o può clamorosamente fallire per dare una risposta seria e adeguata ai problemi che ci vengono proposti dai cittadini. Non credo che sia il caso di mettersi qui a rinfacciarsi o rimpallarsi con gli esponenti dell'antipolitica, o presunta tale, responsabilità, retribuzioni e emolumenti. Credo che la cosa migliore sia quella di dire che l'antipolitica prospera quando la politica non fa bene il suo mestiere, e penso che questa occasione dell'approvazione del bilancio del Senato debba essere quella in cui la politica si riappropria del suo modo di fare bene il proprio mestiere. Il Collegio dei Questori mi consentirà di dire, con rispetto ma anche con fermezza, che il progetto di bilancio che è stato portato oggi alla nostra attenzione è assolutamente inadeguato all'obiettivo che già alcuni interventi hanno proposto; credo anche che se, fino a prima dell'intervento del collega Malan poteva esserci il sentore di poter in qualche modo aggiustare il bilancio che è stato qui presentato con l'approvazione di ordini del giorno (in particolare mi riferisco a quello importantissimo del mio Gruppo parlamentare), mi sembra che, dopo l'intervento del rappresentante del PdL, questa possibilità si sia fatta, a dire il vero, ancora più ristretta.

non si può consentire che tra la mia dichiarazione dei redditi e quella di altri colleghi, senatori o deputati, vi sia un rapporto di uno a sette o di uno a otto, quando il tempo che mettiamo a disposizione della nostra istituzione dovrebbe essere identico.

Voglio fare un esempio. Nel 2001, il fatturato del Senato era di circa 402 milioni di euro,

che, se si vuole davvero affrontare il tema, ai costi della rappresentanza si deve rispondere con un'indicazione netta: quella di portare cioè gli emolumenti complessivi, onnicomprensivi, di senatori e deputati dello Stato italiano alla media europea. Lo abbiamo detto, qui il discorso comincia e qui finisce.

della contabilità industriale, con una riforma profonda dell'organizzazione del Senato e con l'utilizzo pieno del sistema della *spending review*, oppure i responsabili devono applicare una riduzione dei costi che sia comunque di questo ordine. Altrimenti è un gioco, cari colleghi. È un gioco di cui dovremmo rispondere di fronte al Paese, e saremmo noi stessi ad alimentare il clima dell'antipolitica. Passo alla seconda considerazione. Non voglio entrare in questioni su cui hanno già parlato i colleghi e su cui ancora si dirà: a spese che sono assolutamente strepitose e incomprensibili per i più. Come si può spendere tutto quello che si spende per la manutenzione straordinaria degli immobili, che è un importo decisamente superiore al valore degli immobili iscritti nel nostro bilancio? Come si possono spendere 1,5 milioni di euro di facchinaggio, come se noi fossimo tutti impiegati presso la stazione Termini a trasportare colli dalla mattina alla sera?

c'è un certo Luca Pacioli, mio corregionale, che tanti secoli fa - esattamente cinque secoli fa - usò il termine «resa del conto», che non è «Mezzogiorno di fuoco»:

che usano quasi esclusivamente risorse pubbliche, cioè dei contribuenti italiani) deve rendere conto di come usa le proprie risorse. Non mi pare

Mi permetto di dire che, così come si sta ragionando oggi sull'applicazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di stato giuridico dei partiti, si debba parimenti rivedere una certa idea, troppo antica, degli *interna corporis* del Senato.

il tema del bilancio del Senato viene trattato in un momento in cui è in discussione, sui *media* e nel Paese, anche a seguito della crisi economica, la questione dei costi della politica. Automaticamente,

fare di tutta l'erba un fascio. Alcuni interventi sono stati molto puntuali e li ho apprezzati particolarmente, compreso il raffronto con altre istituzioni europee analoghe alla nostra (mi riferisco all'intervento del collega Malan).

Oggi commentavo con un collega la questione del barbiere, che non mi ha mai particolarmente appassionato. Non è un'esigenza che ho sentito molto, almeno da

quel decoro che è fondamentale per rappresentare il Paese, perché il Parlamento è la rappresentanza del Paese. È stato fatto un passo; forse altri possiamo farne su tutta un'altra serie di servizi che riguardano anche il sistema della ristrutturazione e quindi del rapporto con i dipendenti del Senato, o con la gestione degli immobili. È stato previsto di abbandonare alcuni immobili (parlo

deve porselo in proprio per il bilancio del Senato, per i vitalizi e per le indennità dei senatori, ma deve porselo quale legislatore nei confronti di tutto il sistema della politica e delle istituzioni del Paese, stando attenti a distinguere - come dirò - tra partiti e istituzioni, quindi tra gestione della politica e gestione della partitocrazia, cioè il sistema di finanziamento dei partiti. il Parlamento deve stare attento a non avere una funzione demagogica, perché in un momento in cui nel Paese si parla di contratti di solidarietà e poi si legge nella rassegna stampa che la Camera paga per non essere assenti,

inferiore! In questo caso, ho citato quanto ho letto nella rassegna stampa di oggi che riguarda l'altro ramo del Parlamento. Mi auguro che in questo ramo ciò non avvenga,

per adeguare le esigenze al tempo, alle condizioni economiche, alle condizioni sociali e naturalmente, a questo punto, al beneficio e all'alto interesse del Paese che noi dobbiamo perseguire. Quindi, la prima valutazione che lascio al collegio

sono favorevole al finanziamento dei partiti, perché in una democrazia i partiti devono avere un meccanismo di finanziamento e sono

il sistema della politica nelle istituzioni al ruolo e ai carichi che ci sono. C'è un carico sul Parlamento,

noi e prima di tutto il Governo che presenta i provvedimenti, svolgere il nostro compito con un po' più di razionalità e di equilibrio, non sempre con il taglio per emergenza.

manifestano l'incapacità delle democrazie. Chi sostiene il Governo tecnico dichiara che le modalità della democrazia e la rappresentanza politica, peculiare della democrazia,

in secondo luogo, la dignità dei parlamentari che devono onorare con il loro lavoro e non con la loro assenza le istituzioni, perché sono pagati per svolgere il sono pagati per svolgere il loro ruolo, senza però cadere nella codardia di tagliare lo 0,1 perché tutti dicono che dobbiamo tagliare.

per sgombrare il campo da ogni equivoco, vorrei partire da una premessa di metodo e di forma. La premessa di metodo è che ogni singolo euro risparmiato nel bilancio del Senato è cosa santa, giusta e sacrosanta. La premessa l'ho già detto ai senatori Questori in Commissione - è che ritengo assolutamente opportuno, per chiarezza e trasparenza, presentare il bilancio interno del Senato in una sintesi di dieci voci. voci. Dalla sintesi di dieci voci, infatti, si capisce esattamente cosa costa il Senato della Repubblica e perché. Cercherò in questo mio intervento di anticipare i tempi, nella speranza che il prossimo anno il bilancio del Senato venga presentato con questa tabella di sintesi in modo da capire di che cosa stiamo parlando. Ciò detto con queste due premesse, signora Presidente, cari colleghi cari colleghi della maggioranza e dell'opposizione, è indubbio che frequentemente, ogni tre, quattro anni e in questo momento,

che tende ad indicare come costi della politica il bilancio del Senato, il costo dei senatori, il costo delle strutture. Ma è un errore questo? È una non conoscenza? Ho timore di no. Questo polverone mediatico, che concentra l'attenzione su elementi assolutamente irrilevanti dal punto di vista quantitativo, ha come obiettivo quello di nascondere agli occhi dei cittadini i veri costi della politica che non sono misurabili in centinaia di migliaia di euro o in qualche milione di euro dei risparmi fattibili nel bilancio del Senato, ma sono misurati ogni giorno nei dati ufficiali da decine e decine di miliardi di euro malversati, truffati, sottratti alle tasche dei contribuenti onesti e tartassati. E allora, mi permetto di aggiungere alle valutazioni microeconomiche, che condivido totalmente, del collega Malan alcune valutazioni macreconomiche, per capire almeno tra noi di che cosa stiamo parlando. stiamo parlando. Noi politici, maggioranza e opposizione, determiniamo ogni anno 800 miliardi di spesa pubblica. Di questi, 424 miliardi sono decisi al di fuori dell'Aula del Senato e dell'Aula della Camera, perché sono decisi da Regioni, Province e Comuni. Quindi, noi decidiamo ogni anno 376 miliardi di euro di spesa pubblica. di costi della politica, è evidente che dobbiamo andare a vedere con la lente di ingrandimento dentro quelle cifre dove sono i veri costi della politica. A fronte di questi dati, il bilancio del Senato, poco più, poco meno ogni anno, si riferisce a 600 milioni di euro. Tra il bilancio del Senato e ciò che nasconde i costi della politica, cari colleghi, ci sono tre zeri di differenza. Le ruberie e i costi della politica si misurano in miliardi e miliardi di euro; i costi del Senato si misurano in milioni di euro. Ricordo la premessa: ogni euro risparmiato nel bilancio del Senato è cosa sacrosanta. Bene, questi 600 milioni rappresentano lo 0,07 per cento del totale della spesa pubblica, cioè di quella che dovrebbe essere la nostra responsabilità politica di dimostrare ai cittadini come e perché l'abbiamo spesa (si tratta di

di indicare all'opinione pubblica, ma soprattutto il coraggio di tagliare dentro quest'Aula, per decine di miliardi. Vi leggo la tabella ufficiale del Ministero dell'economia: 142 miliardi, chiamati eufemisticamente consumi intermedi, acquisti di beni e servizi. Ci sono dentro almeno 30-40 miliardi di costi della politica, cioè di malversazioni, aree grigie e tangenti, anche con contatti con le grandi organizzazioni criminali. seconda voce, anche se il Ministero dell'economia negli ultimi anni ha tentato di nasconderla, riporta i contributi in conto capitale, che ancora appaiono in modo esplicito in quella tabella ed ammontano a 16 miliardi all'anno, contributi a fondo perduto, costi della politica veri per decine di miliardi, e gli altri 24 miliardi di contributi in conto corrente (da qualche anno non appaiono più esplicitamente perché sono stati nascosti dentro una voce che ha un totale di 61 miliardi di euro, chiamata "Altre uscite correnti"). Questi sono i veri costi della politica. Allora noi abbiamo il dovere e la responsabilità di rispondere ai cittadini italiani per ogni singolo euro di quei 600 milioni spesi per il Senato. La nostra responsabilità vera, però, è di rispondere per ogni singolo euro di quegli 800 miliardi totali o di quei 50-60 miliardi che la Corte dei conti - non solo il sottoscritto, da anni - indica come sprechi, malversazioni e ruberie, cioè costi della politica. Veniamo allora al bilancio del Senato come vorrei leggerlo. Sono circa 600 milioni di euro;

C'è una vera anomalia, cari colleghi, sul sistema pensionistico del Senato - e su questo verte la mia proposta - perché esso è ancora a metodo retributivo.

fatta 16 anni fa? Signora Presidente, dei 400 milioni che costa il Senato, 71 milioni sono gli stipendi dei senatori, 165 milioni sono gli stipendi del personale, 142 milioni è la somma che viene data a supporto dei Gruppi parlamentari; se togliete 22 milioni di partite di giro, abbiamo finito

nascondere agli italiani i veri costi della politica, la non assunzione di responsabilità di quest'Aula nel momento in cui decide il complesso delle spese pubbliche. Chi cavalca quella tigre sappia che, consapevolmente o inconsapevolmente, è complice di chi nasconde agli occhi dei cittadini le altre ruberie per decine di miliardi di euro.

i bilanci, pubblici o privati, sono il documento con il quale ci si presenta all'esterno, si traccia la politica aziendale e si chiedono la fiducia e il consenso alle assemblee. Credo poi che i bilanci si leggano per ciò che dicono, ma molto di più si apprende da ciò che non dicono. Leggerò il bilancio interno del Senato facendo la seguente distinzione: le cose che ho trovato e che mi hanno detto molto, e le cose che non ho trovato, che confesso mi hanno detto di più. due punti fondamentali delle situazioni che ho trovato. Partiamo dall'*incipit* piuttosto impegnativo del bilancio che è stato richiamato anche dal Presidente della Commissione bilancio. Recita l'*incipit* della relazione del bilancio di quest'anno: «Nel contesto della severa manovra di risanamento per il triennio 2011-2013

ineccepibile. Che sacrifici imponeva il decreto-legge n. 78 che abbiamo testé ricordato dello scorso anno? Imponeva delle radicali riduzioni dei costi degli apparati amministrativi, delle pubbliche amministrazioni e del consolidato dello Stato. L'articolo 5, tra l'altro, imponeva a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico della pubblica amministrazione

Rapportato molto "spannometricamente", e per difetto, alla nostra realtà, con esclusione della riduzione dei compensi, che effettivamente sono stati ridotti, nell'ordine del 9,7 per cento - con un piccolo sforzo ci saremmo, quindi, perfettamente adeguati a quanto abbiamo imposto agli altri - per quanto riguarda le altre spese che ho citato, dalle consulenze ai convegni, devo dire che, compresi i sussidi erogati per 1 milione e 350.000 euro direttamente dal Consiglio di Presidenza, ce ne facciamo per un pacchetto da 12 milioni di euro. Se avessimo aderito e partecipato - come detto in premessa - ai sacrifici imposti a tutte le altre amministrazioni inserite nel conto economico della pubblica amministrazione

Quindi, ai tagli che ho richiamato di queste voci oggettivamente comprimibili, sono stati obbligati dall'Agenzia spaziale all'ENEA, dal CNR alla Lega tumori, dalla Triennale di Milano all'INPS: certo, obbligati sotto la mannaia della responsabilità disciplinare ed erariale. Perché non il Parlamento della Repubblica? Non l'ho capito e avevo presentato un emendamento in tal senso, che è stato ovviamente respinto, e credo di non essermi fatta neanche degli amici, ma si tratta di un dato irrilevante. Ce ne sarebbe stato bisogno? Credo proprio di sì. È stato ricordato dai colleghi che mi hanno preceduto un dato che parla da solo: in dieci anni il costo del Senato è aumentato di 200 milioni di euro, per cento in più in dieci anni. Direi che è un costo oggettivamente da monitorare. Ricordo, per inciso, che la spesa per le indennità, invece, è scesa, in questo stesso decennio, di

Questo dato, che ha scatenato anche applausi, convince, ma soprattutto temo che convinca più noi che il resto del mondo. Quindi, siamo compiaciuti di essere in adeguata compagnia, e non troppo lontani dagli altri, ma questo non ci avvicina al resto del Paese, né ci fa superare il problema che tutti hanno prima rilevato, vale a dire la pesante cappa di

E temo che non stia funzionando l'azienda Paese, e sono certa che non sta funzionando l'azienda Senato, per le ragioni che ho detto. Un'altra voce che trovo scritta nel bilancio del Senato riguarda le spese di personale: altra voce assolutamente rilevante. Trovo scritto, tra le politiche del personale,

Veniamo alla prima voce: razionalizzazione. Ho cercato riscontro nei numeri e all'interno del bilancio: io non trovo una traccia di riorganizzazione. Non trovo traccia di eliminazione di servizi obsoleti, e mi affanno a dire, quale disturbatore di Assemblea, tutte le volte che approviamo il bilancio, che non capisco perché in Senato si entri da cinque porte, di cui quattro ampiamente presidiate; che non capisco perché nel Senato della Repubblica debba esserci un guardaroba che, soprattutto nella stagione estiva, non ha ragione di esistere, perché non c'è niente da guardare, e il problema potrebbe benissimo essere diversamente risolto; non capisco perché debbono esserci guardianie con decine di persone ai piani, quando con un *badge* avremmo accesso agli uffici. E ripeto, come un disturbatore di Assemblea a ogni approvazione di bilancio, non ho avuto la grazia di una risposta e non trovo qui la traccia di un'iniziativa.

Io credo che l'alto costo del personale del Senato sia legato al fatto oggettivo dell'alta qualificazione del personale del Senato, ad ogni livello. Di norma, in nessuna azienda si rende compatibile l'alta qualificazione con la consulenza, soprattutto a questi livelli. Può essere anche necessaria qualche consulenza specifica, ma spendere 140 milioni di euro per il personale dipendente e poi ricorrere a 6.300.000 euro per le consulenze, mi sembra un dato difficile da tener insieme. poi sottolineare, in particolare rispetto ai tagli di spesa sul personale che si sarebbero fatti, un dato molto significativo su cui richiamo l'attenzione della Presidenza, dei signori Questori e dei colleghi senatori. Noi abbiamo letto che sono contenuti i costi di personale. In verità, il costo del personale complessivo del Senato, costituito da personale dipendente, non dipendente e da personale dei Gruppi, ammonta oggi a 178.800.000 euro, 250.000 euro in più rispetto al 2010:

14 milioni di euro. Complessivamente, siamo a 178.800.000 euro. Questo vuole anche dire che, mentre sta diminuendo il personale dipendente del Senato, e può essere una logica politica di contenimento che porterà, insieme a tante ristrutturazioni che spero ci saranno, a un contenimento dei costi,

della Costituzione, che prevede: "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione". I pubblici I pubblici impiegati, infatti, sono esclusivamente al servizio della Nazione. Devo però dire che, quando il personale non è dipendente, viene scelto discrezionalmente e senza concorso, il principio

delle istituzioni, fanno fatica a sostituire il messo comunale. Passiamo quindi, e molto rapidamente, a ciò che il bilancio non dice. Non dice cosa e come si intenda razionalizzare. Li ho ricordati prima e non sto certo a ripeterli adesso, certo a ripeterli adesso, ma alcuni costi, che vanno dai supporti informatici per il mandato dei senatori, che vedo riportati ogni anno in cifra considerevole e che poco giustifico, alle notevoli spese per l'ordinaria amministrazione,

molto mi dispiaccio. Non c'è la leggibilità reale del bilancio. Non c'è la distinzione tra il patrimonio del re e il patrimonio dello Stato. E se dovessi dire, scendendo di molto rispetto a ciò che non c'è, non c'è neanche chi rilegga le carte e dia qualche pietoso tratto di penna, sia sui refusi tecnici sia sui refusi d'immagine. Mi riferisco ai 40.000 euro di posate, che credo annualmente non sia il caso di spendere.

In realtà, i cittadini, quando hanno votato contro quella riforma costituzionale, non si sognavano neanche per caso di votare contro la riduzione del numero dei parlamentari. Hanno votato contro una forzatura della Carta costituzionale in senso fortemente presidenzialista, con un rafforzamento dell'Esecutivo, un abbattimento delle potestà degli altri poteri e una distorsione dei rapporti tra il potere esecutivo e la magistratura. Se i cittadini avessero potuto votare soltanto la riduzione del numero dei parlamentari, l'avrebbero fatto gioiosamente, solo che voi non avete dato loro questa possibilità. alla questione dei costi della politica. Voglio chiamare in causa un convitato di pietra, che non ci compete in questo momento, ma che sono costretto a ricordare. È vero che le Camere costano moltissimo, ma che dire della voragine incalcolabile dei costi che la Presidenza del Consiglio si porta dietro di sé, con l'attribuzione delle spese per la Protezione civile, la gestione dei grandi eventi?

di far lavorare le Camere anche ad agosto. Penso che se davvero, lavorando in agosto, si continuassero a produrre nefandezze come quella sul "processo lungo", sarebbe molto meglio andare in vacanza. In fondo, l'esempio del Belgio, un Paese che, pur senza Governo da più di un anno, riesce a resistere, dimostra che potremmo benissimo fare a meno del Governo Berlusconi.

Tutti noi sappiamo che, per i collaboratori, i senatori percepiscono un po' più di 4.000 euro al mese. Spendono davvero questa cifra per i collaboratori? No.

un dato certo, sulla Camera sappiamo che i collaboratori sono 230. Questo significa che ci sono circa 400 deputati che non hanno un collaboratore o, se lo hanno, non ce lo fanno sapere; quindi, si spendono un sacco di soldi

di 4.000 euro al mese al Senato stesso, senza passare attraverso i senatori. Questa cifra sarà spesa soltanto nei casi in cui sarà dimostrato

Non so fare il conto di quanto si potrebbe risparmiare, però sta alla vostra intuizione ragionarci sopra, facendo un rapido conto di quanti sono i senatori che non dichiarano apertamente un rapporto con un collaboratore. In più, ciò garantirebbe una notevole trasparenza, perché il collaboratore avrebbe un rapporto diretto con la Camera elettiva e il senatore non potrebbe intascare, come fa ora, una parte del contributo che riceve perché non lo percepirà nemmeno. Quei soldi passeranno, infatti, attraverso un altro circuito, e la situazione sarà molto più chiara e trasparente. In questa maniera eviteremmo di accumulare ragioni perché si possa parlare - e questa volta a ragione delle nostre mancanze e stabiliremmo un criterio estremamente pulito e privo di possibilità di imbroglio per la remunerazione del prezioso lavoro dei collaboratori. Ricordo infine che questa maniera un po' truffaldina di trattare i collaboratori, pagandoli e non pagandoli - sono note tra noi le storie di molti senatori che pagano in nero dei collaboratori schiavizzati

non piace a molti colleghi. So che si rischia l'ingenuità a sostenere queste cause. Si fa la parte di quelli che sono stati paracadutati in un mondo che non conoscono e che ignorano le regole nascoste del vivere qui dentro. non me ne importa niente. Secondo me, la proposta ha una sua chiarezza, ha un significato di pulizia e anche di impegno nei di impegno nei confronti dell'opinione pubblica. Facciamo penetrare lo sguardo dei cittadini in queste cose. Esponiamoci. Il Parlamento deve essere una casa di vetro. Smettiamo di nascondere le nostre cose. Mettiamoci di fronte al giudizio dei cittadini, e vedrete che alla fine anche la nobiltà della Camera elettiva ne trarrà un vantaggio significativo. Signora Presidente, il 22 giugno scorso ho già avuto occasione di attirare l'attenzione del Senato sulla anomalia originata da una delibera della Presidenza del Senato stesso del 1993 e da alcune altre delibere analoghe, che si sono succedute all'inizio di ciascuna legislatura, in materia di personale dipendente dai Gruppi. Credo sia necessario tornare su questo argomento per il rilievo che esso assume in sede di bilancio del Senato, per sottolineare l'ingiustizia che da questo assetto consegue quotidianamente tra queste mura tra i dipendenti dei Gruppi e, se possibile, per indicare un modo in cui - a mio avviso - questa ingiustizia e questa anomalia possono e debbono essere eliminate. Da molti anni, analogamente a quanto avviene alla Camera dei deputati, in tutti i Gruppi parlamentari si è determinata una situazione di marcata differenza di trattamento tra i dipendenti assunti sulla base della delibera - cui accennavo - del 1993 o di altre successive, volte a favorire l'assorbimento dei dipendenti dei Gruppi estinti da parte dei Gruppi attivi, dei Gruppi attivi, e i dipendenti non assunti sulla base di quei provvedimenti. I primi sono assunti a tempo indeterminato con un trattamento mediamente molto più alto rispetto ai secondi, i quali sono assunti a termine, talvolta addirittura con rapporto di lavoro a progetto, e si vedono riservare, anche a parità di mansioni o addirittura svolgendo mansioni professionalmente molto più qualificate, un trattamento mediamente molto più esiguo. Il progetto di bilancio che ci è stato presentato prevede a questo proposito due contributi del Senato ai Gruppi, che compaiono nel capitolo S.1.08: il primo, come contributo proporzionale alle dimensioni dei Gruppi; il secondo, consistente in rimborsi forfetari per i dipendenti assunti in base alle delibere che ho menzionato. La prima questione che intendo proporre riguarda proprio questo capitolo del bilancio. Logica e rispetto del Regolamento del Senato vorrebbero che i due contributi in esso previsti venissero accorpati in un contributo unico, proporzionato alle dimensioni di ciascun Gruppo. Questo anche per ricondurre l'intero capitolo alla piena trasparenza che, con l'istituzione del contributo forfetario, è andata perduta, poiché nessuno sa né può leggere nel bilancio dove vadano quei 12 milioni: erano 11,9 nel 2010 e adesso addirittura sono aumentati a 14 milioni.

mediamente utilizzato soltanto per due terzi per la copertura dei costi dei rapporti di lavoro costituiti in base a quelle delibere; il terzo mediamente restante costituisce una differenza che il Gruppo datore di lavoro incassa in aggiunta al contributo ordinario di cui alla prima voce del capitolo in esame. Ho verificato che, anche a spesa complessiva invariata per il Senato, l'operazione di accorpamento di questo contributo con l'altro e il riproporzionamento complessivo del nuovo contributo unico alle dimensioni dei Gruppi può avvenire incidendo soltanto sulla differenza incamerata dal Gruppo e senza che venga intaccata la parte del contributo che serve effettivamente a coprire il costo dei rapporti di lavoro, così come oggi distribuiti. Quindi, l'accorpamento dei due contributi e il riproporzionamento complessivo degli stessi può essere attuato anche senza cambiare di un euro il trattamento dei dipendenti assunti in base alle delibere, se è questo che si decide di fare. Resta però una seconda questione (connessa a questa, ma concettualmente distinta) che concerne l'assetto giuridico ed economico dei rapporti tra i Gruppi e i rispettivi dipendenti. Menziono questo problema non perché esso possa essere risolto in sede di approvazione del bilancio del Senato, ma perché credo che nella decisione sulla prima questione la Presidenza del Senato debba anche porsi il problema di incentivare

tutti i rapporti di lavoro, sia quelli costituiti in base a delibera sia quelli non costituiti in base a delibera, sono rapporti di natura privatistica che non comportano alcun rapporto contrattuale o di altro genere tra il lavoratore e il Senato. Nulla impedirebbe dunque che ciascun Gruppo procedesse a un riordino generale dei trattamenti per parificare innanzi tutto il tipo di contratto;

potrebbero benissimo essere assunti tutti a tempo indeterminato con previsione esplicita del recesso all'inizio della nuova legislatura in caso di riduzione degli organici o cessazione dell'esistenza del Gruppo,

Occorre poi istituire un sistema di inquadramento professionale degno di questo nome; e vorrei ricordare a questo proposito che l'obbligo

parità di trattamento. Non è possibile stabilire parità di trattamento a parità di mansioni se non c'è un criterio di valutazione delle mansioni. un sistema di inquadramento che consenta di individuare il trattamento riservato a ciascuna categoria e qualifica; questo consentirà di chiarire c'è qualche dipendente fortunato, assunto in base a delibera, che gode di un superminimo *ad personam*, beneficio economico che quindi verrà individuato come tale e che potrà essere assorbito nelle dinamiche economiche successive. Ma se non cominciamo a compiere quest'opera, questo assorbimento progressivo non avverrà e la disparità di trattamento andrà aggravandosi, invece che ridursi, per effetto delle dinamiche di anzianità. Tutto ciò secondo una prima soluzione possibile,

comportando una almeno parziale redistribuzione dell'enorme differenza di retribuzione che oggi distingue tra loro anche persone che fanno esattamente lo stesso lavoro, differenza che privilegia assurdamente persone che svolgono un lavoro di livello nettamente inferiore rispetto a quello di altre che ne svolgono uno molto qualificato. Poiché le retribuzioni di cui godono gli assunti in base a delibera sono di molto superiori a qualsiasi possibile standard inderogabile di riferimento, nulla vieterebbe alle parti di rinegoziarle con con previsione di una loro riduzione, magari di modesta entità, in funzione di un corrispondente aumento delle altre; una pattuizione di questo genere sarebbe perfettamente valida ed efficace.

per incentivare una razionalizzazione su questo terreno. Le delibere che ho menzionato all'inizio e che si sono succedute dal 1993 in poi non hanno più alcuna ragione d'essere oggi servono soltanto come fonte dell'impegno per il Senato di corrispondere ai Gruppi il rimborso forfetario, che deve essere invece incorporato nel nuovo contributo unico proporzionato alle dimensioni dei Gruppi. Per questo motivo l'ordine del giorno G5, che reca la mia prima firma insieme a quella di altri colleghi, si propone di voltare pagina rispetto alla stagione di quelle delibere. Da parte di diversi colleghi, anche investiti di responsabilità di gestione in questa istituzione, ci è stata rivolta la richiesta di ritirare quell'ordine del giorno, per consentire un approfondimento delle questioni, certo non semplici, implicate in questo disegno. Accogliamo questa richiesta, per dar modo a tutti gli organi del Senato, a cominciare dalla Presidenza e dal Collegio dei Questori, di studiare più attentamente le questioni proposte; molto più attentamente di quanto non risulti da questo progetto di bilancio, nonostante che le questioni stesse siano state già poste nel mio intervento in quest'Aula del 22 giugno scorso. Mi auguro, anche per l'onorabilità sostanziale della nostra istituzione, che prima della fine di quest'anno sappiamo voltare pagina definitivamente rispetto alle opacità, alle rendite indebite e alle irragionevoli disparità di trattamento che dal 1993 in poi quelle delibere hanno generato. Terzo Polo:ApI-FLI)*. Signora Presidente, l'esame del bilancio del Senato della Repubblica per l'anno 2011 è accompagnato da numerose suggestioni endogene ed esogene. Tra le prime, segnalo l'ansia da comunicazione per la quale conta chi arriva primo a dire qualcosa, piuttosto che l'oggetto comunicato. Penso alla gara - mi consenta di dire - ridicola tra Senato e Camera a dire chi taglia di più e chi lo fa prima. Sono iniziative che cercano di venire incontro ad una sete di giustizia istituzionale che proviene da tutta Italia, ma che finiscono con il peggiorare l'immagine del Parlamento. Più che parole, occorrono fatti, e comunque le une e gli altri vanno proposti con franchezza e precisione, senza ipocrisie, infingimenti o arroganze. A proposito di parole, sono rimasto colpito da un passaggio del discorso del nostro Presidente

(si riferiva esplicitamente alla documentazione depositata per la nota vicenda del senatore Tedesco). Non mi è parsa una cortesia del signor Presidente nei nostri confronti. Proprio in quest'Aula, pochi giorni fa, un autorevole Ministro del Governo provvisoriamente in carica ci ha ricordato che, in caso di naufragio, ci si inabissa tutti. Mi aspetterei le scuse del Presidente per quella sua frase. Tant'è, il vizio di dare pagelle è esteso. Giorni addietro è capitato pure ad uno stimabile collega di tracciare una sorta di profilo del senatore, salvando gli accademici e dannando come nullafacenti tutti gli altri. Credo che dovremmo tutti, piuttosto, avere a cuore la dimensione politico-istituzionale e, in questo senso, la dignità del nostro ruolo, recuperando al nostro interno anche il necessario mutuo rispetto, che la capacità e la sapienza pedagogica di presentare efficacemente il Senato della Repubblica nelle sue funzioni costituzionali come un baluardo della democrazia. Nelle ubertose convalli trentine dalle quali provengo, i vigneti producono quantità straordinarie di ottima uva, dalla quale vengono ricavati vini spesso pregevoli: alcuni godono della denominazione di origine controllata (DOC) e sono infatti imbottigliati e presentati conseguentemente; altri si vendono in bottiglie standardizzate, il cosiddetto tappo a corona. Ecco, anche fra i senatori c'è il DOC e il tappo a corona: ma sempre senatori siamo. Se ci rispettassimo reciprocamente un po' di più, l'immagine - per quello che conta - ne risulterebbe valorizzata. Rappresentiamo l'Italia e mediamente la cosiddetta società civile - dalla quale peraltro proveniamo - è esattamente qui in mezzo a noi descritta. Certo, dall'esterno provengono poi ben altre suggestioni: casta è termine ormai gergale per indicare i politici in genere e i parlamentari in particolare, ed è innegabile che la letteratura in merito possa attingere a circostanze, fatti e vicende assolutamente non confacenti al ruolo che tutti noi temporaneamente impegnati in politica dovremmo positivamente assolvere. Non mi riferisco solo alle palesi illegalità per le quali la giustizia deve fare sempre il suo corso; mi riferisco, piuttosto, a quella immensa palude di contaminazioni di interessi, di leggerezze, di menzogne e di favoritismi nella quale risultano effettivamente coinvolti molti - forse troppi - di coloro che finiscono per questo nel mirino di giornali e di commentatori. Per evitare che la somma di queste suggestioni endogene ed esogene possa condizionare le nostre odierne riflessioni nel nome troppo facile dell'antipolitica, o nell'invito già risuonato a non abbandonarsi alla facile demagogia, forse è il caso di tentare un approccio assolutamente concreto al bilancio in esame, chiedendoci se l'orientamento vada nel senso di qualificare ruoli e funzioni; se le scelte sulla prospettiva della sobrietà e del risparmio, quanto mai coerenti con le difficoltà dell'ora, siano sufficienti e soprattutto comprensibili; se, ed eventualmente dove e come, sia possibile fare di più.

La spesa pubblica va ridotta e, in questo senso, anche il Senato della Repubblica fa la sua parte. Sull'effettiva declinazione di tale opzione, tuttavia, esprimo il dubbio che si sarebbero potute compiere scelte ben più incisive, direttamente connesse anche ad un cambio di approccio politico e culturale al nostro cosiddetto *status* e all'invalso modello organizzativo interno. Occorrerebbe tuttavia, per questo, una palese espressione di volontà da parte dei diversi Gruppi, o almeno da parte dei loro vertici. la vicenda raccontata in Aula poco tempo fa, e ripresa oggi dallo stesso senatore Ichino, su quote di personale fantasma, pagato dal Senato e gestito anche *extra moenia,* è piuttosto grave. Certo, c'è un ordine giorno in merito (che ho sentito poco fa che verrà ritirato), ma penso che Questori e Consiglio di Presidenza dovrebbero già aver assunto drastiche decisioni in proposito, con palesi ulteriori risparmi. Per quanto riguarda le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori, dall'intemerata a regolarizzare i rapporti di lavoro (evidentemente lanciata per chi non era in regola), corredata da scadenze temporali e sanzioni operative, è passato un anno e non sappiamo gli esiti. Forse qualche senatore paga in nero il proprio collaboratore? Non credo ci voglia molto per fare ordine nello specifico. Sulle cosiddette auto blu, oggetto di una precisa norma della recente manovra, quale orientamento si intende assumere? Leggo in relazione che si cerca una sede per l'autorimessa. le auto di servizio del Senato? Chi ne usufruisce? Qualcuno può rinunciare a favore di *taxi* o mezzi pubblici? Non è demagogia: come diceva il collega Giaretta, si tratta di scegliere un modello di stare nelle istituzioni e di contribuire a caratterizzarle.

della ristorazione. Perché non fare come per la barbieria? Aperta sì, ma a prezzi di mercato. C'è già una voce sui rimborsi spese che calza esattamente sui costi della nostra settimanale presenza romana. Può essere utilizzata anche per i pasti, realizzando un notevolissimo risparmio per il bilancio del Senato.

Non sarebbe ora di togliere di mezzo questo beneficio, come ogni altro beneficio eventualmente riconosciuto agli ex? Ricordo che fra poco noi saremo tra gli ex. A ricordo dello *status* restano il titolo e, da una certa età, il vitalizio. Proviamo a dire oggi che può bastare: anche in questo caso, senza demagogie, ma per delineare piuttosto un modo diverso di rapportarci alle istituzioni. Nessuno può contestare un'indennità importante ai parlamentari che, nello svolgere il loro compito, devono essere cittadine e cittadini assolutamente liberi da condizionamenti. diversi *extra:* gli sconti per servizi, le facilitazioni per teatri, stadi, viaggi e quant'altro (nel quant'altro segnalo gli alloggi di servizio, della cui esistenza apprendo dalle cronache, che sarebbero disponibili per alcune categorie di senatori: mi chiedo se sia vero e se non sia possibile eliminare tale voce). Gli *extra* e il permanere di parti di essi dopo il mandato sono elementi che, prima ancora che dalla forte sensibilità sociale oggi emergente, dovrebbero essere considerati esuberanti da noi stessi e da coloro che in questo ruolo ci hanno preceduti: una sobrietà non forzata, ma coerente con lo stile di vita della maggioranza di noi parlamentari. Credo non basti la personale rinuncia a questo o a quello o la devoluzione in beneficenza. Trattandosi di denaro pubblico, la scelta dovrebbe essere politica e in radice: si taglia per tutti. Così, credo ci sia spazio nel nostro bilancio anche per qualche ulteriore riduzione nella manutenzione e negli acquisti (capitoli 1.24, 1.25, 2.30, 2.31). Ma vi paiono sensate le corsie rosse sulle scale del cosiddetto ex Bologna? Ci sono anche altri temi, ai quali accenno solamente, e concludo, signora Presidente. Mi ha sempre appassionato, in questi anni, l'analisi del nostro bilancio compiuta dal collega Morando e la sua proposta di coordinare i Servizi bilancio di Camera e Senato. Se ho capito bene dalla relazione, siamo in proposito ancora alle lontane premesse. È possibile accelerare? E ancora: a cosa è dovuta l'esplosione dei costi, ricordata da tanti in questa sede, per il personale addetto alle segreterie particolari (più un milione e mezzo di euro, cioè più 11 per cento)? Si potrebbe avere un dettaglio della voce? Infine, signora Presidente, si apprende dalla relazione che i Questori e il Consiglio di Presidenza, volendo dare positiva risposta alla recente manovra nell'articolo che riguarda le nostre indennità complessive, intendono avanzare una proposta di riordino delle indennità, e spero anche in una rivisitazione del tema vitalizi. Mi parrebbe di buon senso, in tale contesto, al fine di favorire la qualità del nostro lavoro e di mettere a tacere le malelingue, prevedere che anche l'assenza dai lavori delle Commissioni permanenti e delle bicamerali sia sanzionata in busta a fine mese. È un modo un po' forzoso, se vogliamo, per migliorare la nostra produttività sempre a beneficio del Paese. Con attenzione ai temi proposti, in attesa delle delucidazioni richieste, mi riservo il voto su questo provvedimento.

quello più sbagliato sia quello che consiste nell'approccio meramente contabilistico al problema del bilancio. Opterei, fra le tante soluzioni alternative, per una visione più neosistematica, tipica di chi guarda l'albero senza perdere di vista il bosco. Da questo punto di vista, l'intervento del senatore Malan, che ho condiviso quasi integralmente per i primi due terzi, ha avuto, a mio parere (quindi è soggettivo), una caduta di stile - niente di più - nel momento in cui, invece di continuare sulla giusta linea di ricordare la verità dei fatti, a scapito della inutile demagogia con la quale ogni giorno ciascuno di noi si trova a fare i conti, si è avviato su un cammino - sul quale non lo seguirò - che ha riguardato un attacco ad una parte di questo Parlamento.

perché nessuno di noi può affrontare questo problema pensando che sia sufficiente un inutile esercizio di autodifesa. Io odio il termine casta: mi dispiace anche che un ex collega del nostro Gruppo abbia scritto un libro, insieme ad altri, citando spesso questo termine, però, questo inutile esercizio di autodifesa è esattamente quello che più ci danneggia, non ci aiuta. Mi piacerebbe che una volta il senatore Malan, dietro un vetro che lo oscura (lo richiamo soltanto perché utilizzo strumentalmente il suo intervento, collega, non per polemizzare), partecipasse ad una delle nostre assemblee (nostre, non vostre), dove noi andiamo a spiegare quello che facciamo su questa materia, all'indomani o prima della manovra della settimana scorsa, dove spieghiamo le cose come stanno e come le stiamo gestendo. La risposta sarebbe, alla fine dei due terzi dell'intervento del va bene, insomma ci volete dire che siete poveri, che state morendo di fame! Questa è la risposta che viene fuori da quest'Aula, collega Malan, se lei approccia il discorso in quel modo. Infatti, lei non ha detto falsità; lei ha fatto un elenco onesto e corretto dal punto di vista intellettuale di quello che accade, ma fuori da queste Aule c'è un problema diverso da gestire: per un verso si chiama credibilità, per un altro si chiama onorabilità e per un altro autorevolezza. Scelga lei. È un po' come la questione a tutti nota della sospensione dell'adeguamento dell'indennità parlamentare prevista nella legge finanziaria a far data dal 1° gennaio 2008, che noi abbiamo fatto - noi, non ho detto il Governo Prodi, perché l'avete votato anche voi eppure nessuno lo sa, oppure nessuno lo dice. Anche se se ne parlasse, comunque, non avrebbe lo stesso valore, a fronte di un soggetto molto più autorevole che oggi lo sta facendo, e che è il Presidente della Repubblica. Molto più autorevole significa che quel soggetto ha oggi un'*audience*, viene ascoltato: noi, se diciamo le cose come stanno, rischiamo di non essere ascoltati, per essere diplomatici. Signori Questori, voi avete presentato un bilancio che taglia lo 0,34 per cento della spesa complessiva.

Non sono tirati a "capocchia": spero che qualcuno possa, senza offesa, attribuire a molti di noi che stanno intervenendo alcune competenze, e mi fermo qua. Non parlo delle manutenzioni straordinarie, i cui costi ogni anno hanno bisogno di lievitare progressivamente e necessariamente; non parlo delle manutenzioni ordinarie, sulle quali si aumenta almeno l'indice d'inflazione. Parlo di una serie di cose che fuori di qui non si spiegano: parlo delle segreterie particolari, delle prestazioni professionali, delle consulenze di Commissioni e Giunta, dei Gruppi parlamentari, dei servizi televisivi, delle multimedialità, del personale dei Gruppi che è in carico al Senato, delle locazioni, delle manutenzioni ordinarie agli impianti di sicurezza (con lo *spread* in più dell'aggiunta determinata dall'aumento del tasso d'inflazione per l'anno), della manutenzione per condizionatori, delle imposte, degli impianti che sono stati utilizzati, della rete informatica, del fondo di parte corrente e degli acquisti audio-video. Sapete cosa ho citato? Capitoli sui quali avete apposto aggiunte rispetto all'anno passato. Non sto parlando, infatti, del consuntivo, che non discuto nemmeno, e che do per approvato personalmente e presuntuosamente,

abbondantemente sopra lo 0,34 per cento. Cambio argomento perché i minuti sono pochi. Nel 2007 venimmo sbeffeggiati da una parte di quest'Aula, perché 40 senatori inviarono al presidente Marini e al Consiglio di Presidenza, dove tutti sono rappresentati, un sistema di riordino dei vitalizi parlamentari - il primo firmatario era un certo Luigi Lusi, ma c'erano 40 senatori di molte forze politiche - che applicava immediatamente il sistema contributivo e creava di fatto un'operazione che, portata a regime, avrebbe fatto risparmiare al Paese e ai contribuenti molti denari da allora. Ce la cavammo con qualcosa che era meglio della fotografia di allora, ma non abbastanza, tanto è vero che a distanza di quattro anni è di questo che stiamo parlando. Ce la cavammo con alcune cose che il collega senatore Questore anziano

Noi abbiamo bisogno di subire la critica esterna per avere necessità di trovare risposte, invece di essere noi fautori di una proposta diversa e nuova. È qui che viene in tutta la sua forza l'importanza ed il ruolo dei senatori

nel sistema europeo - quindi non in casa nostra, di cui parliamo sempre male - esiste, oltre alla certificazione dei bilanci, soprattutto un lavoro che è fatto dai revisori del Parlamento stesso; esistono le giustificazioni delle spese;

Mi chiedo: perché alcune Commissioni usano gli aerei di Stato? Perché non volano con Alitalia? Perché non operano con i sistemi normali? Qualcuno mi vuole per caso dire che il costo effettivo, proporzionato all'utente dello Stato che sale sull'aereo di Stato, è inferiore al costo di Alitalia? Prima me lo dimostrate e poi chiedo scusa. Ma come mai? Io, Io, quando l'ho scoperto, sono rimasto allibito. Vi prego di non rispondermi che gli aerei di Stato sono a carico della Presidenza del Consiglio. Risparmiatemi questa rispostina. So che voi tre non me la darete: l'ho anticipata io, e vi ringrazio della cortesia. Ma è un segnale evidente, Presidente, di certe situazioni.

Credo sia importante fare una brevissima sintesi del contesto nel quale oggi svolgiamo questo dibattito sul rendiconto delle entrate e delle spese del Senato e sul progetto di bilancio per l'anno finanziario 2011. Presidente, non al contesto della pressione dell'opinione pubblica e della situazione che vede il Paese impegnato in un incalzante dibattito sul risparmio delle spese,

Un percorso di risanamento che ha visto il nostro Paese sempre più inserito all'interno di un quadro comunitario; l'Italia è stata infatti uno tra i primi e più solerti Paesi ad adeguarsi alle regole del Semestre europeo. europeo. Questo percorso è noto a tutti, naturalmente con differenzazioni sui commenti e sulle valutazioni rispetto alle azioni intraprese dal Governo. Non è possibile negare e contestare il fatto che, per quanto riguarda gli obiettivi più all'attenzione dell'Unione europea, riguardanti il contenimento delle dinamiche del deficit

Queste misure naturalmente hanno richiesto tagli e sacrifici ad una grandissima parte del Paese, alle più importanti istituzioni, alle imprese ed ai cittadini.

in legge il risparmio delle spese delle istituzioni più importanti del Paese, a cominciare dagli enti locali periferici

si era adeguata a queste norme nel rispetto della propria autonomia che - senatore Agostini - ritengo sia una caratteristica irrinunciabile per un Parlamento di uno Stato democratico. Sono favorevole alle ipotesi di revisione dei bilanci e di una commissione interna, ma non credo che possiamo saggiamente rinunciare all'autonomia del Parlamento - perché sarebbe gravissimo - anche sulle questioni che riguardano i propri bilanci. Come è stato detto anche dai colleghi che mi hanno preceduto, già dall'inizio di questo millennio, da dieci anni a questa parte, c'è stato uno sforzo di contenimento dei costi della struttura. In particolare, questo sforzo si è concentrato, un po' per pressione dell'opinione pubblica e un po' per senso di responsabilità - i dati li ha tra gli altri, anche il senatore Agostini - sulle spese della rappresentanza, sulle spese delle nostre indennità che, rispetto al totale delle spese della struttura, sono - come è stato già ampiamente e nel dettaglio illustrato - di molto diminuite, in particolare dal 2001 ad oggi. È questo il contesto in cui noi stiamo affrontando questo dibattito, che ritengo, la ricchezza degli interventi, per il loro dettaglio, per la capacità di esprimere le varie posizioni di entrare nei dettagli delle poste, anche un grande segno di trasparenza che oggi

di contenimento della spesa del Senato, che si è concretizzato nei documenti di bilancio che i senatori Questori hanno predisposto. In particolare - come è stato già detto - ammontano a 120 milioni di euro i tagli alle spese del Senato nel periodo 2011-2014, cifra che comprende i 58,7 milioni di risparmio nel triennio 2011-2013, già decisi nei mesi scorsi e che davano seguito alle previsioni del del 2010, e i 61,3 milioni di euro derivanti dai più recenti interventi; considerato che si è data puntuale applicazione alle misure previste dal decreto-legge n. 98 del 2011 al contributo di perequazione del 5 e del 10 per cento sui vitalizi degli ex parlamentari e sulle pensioni dei dipendenti che superano, rispettivamente, i 90.000 e i 150.000 euro, che già nel 2011 recherà nelle casse dello Stato 1,1 milioni di risparmi, che raggiungeranno 102,7 milioni nel 2012, 2,9 milioni nel 2013 e 3,2 milioni nel 2014. Dopo i tagli alle retribuzioni più elevate, già in vigore dal gennaio 2011, il blocco dell'adeguamento dell'indennità e dei vitalizi dei senatori, nonché il prolungamento al 2014 del taglio delle competenze accessorie ed una serie di ulteriori risparmi, comporteranno una riduzione complessiva della spesa di circa 14 milioni di euro di circa 14 milioni di euro nel biennio 2013-2014; considerato che ulteriori risparmi per 2 milioni di euro deriveranno dallo spostamento del magazzino generale, attualmente collocato nella sede del Trullo,

i tagli sui contratti di utenza per circa 1 milione di euro; considerato che il Senato risparmierà rispetto alla Camera circa 10 milioni di euro in quanto i dipendenti non riceveranno l'aumento del 3,2 per cento sulle retribuzioni riconosciuto nei giorni scorsi al personale di Montecitorio in cambio di nuove norme antiassenteismo, che a Palazzo Madama sono in vigore già da tempo e in forma più restrittiva; ed impegna il Collegio dei Senatori Questori ed il Consiglio di Presidenza: a mantenere invariata nel triennio la dotazione ordinaria (che, per il Senato, costituisce di gran lunga la principale entrata), in modo da assicurare al bilancio dello Stato un considerevole risparmio e delineare con rigore l'entità delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno interno; a valutare la possibilità di redigere un documento finanziario di accompagnamento del bilancio annuale che, traguardando un orizzonte temporale di legislatura, contenga una programmazione funzionale delle spese e degli interventi da effettuare, per non avere come unico riferimento la spesa storica, ma concentrarsi anche sugli obiettivi delle singole poste di bilancio; ad apportare allo stesso strumento di bilancio quelle modifiche espositive che consentano una ancora maggiore trasparenza, anche attraverso informative più dettagliate delle singole poste, mettendo in adeguata evidenza le spese direttamente connesse al funzionamento dell'istituzione e a rendere la documentazione ancor più facilmente consultabile all'interno dei siti Internet del Senato;

a prevedere, d'intesa con la Camera dei deputati, ulteriori interventi volti a dare autonoma attuazione ad altri indirizzi di contenimento della spesa, mirati in particolare a a realizzare, contestualmente alla revisione dell'indennità parlamentare di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 98 del 2011, un riordino delle competenze accessorie ed una riforma della disciplina degli assegni vitalizi, nonché, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, una limitazione nel tempo dei benefici che vengono riconosciuti ai Presidenti dopo la cessazione dalla carica, anche attraverso iniziative iniziative tra i Presidenti del Senato, della Camera dei deputati e della Corte costituzionale; a proseguire nel blocco del *turnover* selettivo del personale, mirando ad una progressiva riduzione della consistenza numerica dell'organico, associata ad adeguati interventi di riorganizzazione funzionale della struttura e, ferma restando l'applicazione del metodo contributivo già vigente per il calcolo dei trattamenti pensionistici, a introdurre anche idonee forme contrattuali da applicare a nuove figure professionali più rispondenti alle mutate esigenze di funzionamento dell'amministrazione; a prevedere, e credo che sia un punto qualificante, che vengano perseguite, previa intesa tra le rispettive Presidenze,

corso dell'approvazione della legge di contabilità), al fine di evitare duplicazioni e favorire sinergie e risparmi nelle aree di supporto documentale all'attività parlamentare, quali ad esempio i Servizi del bilancio, del bilancio, studi e biblioteca; a proseguire, infine, nel percorso di razionalizzazione della complessiva politica immobiliare, che si è avviato con la disdetta della locazione dell'ex hotel Bologna e del magazzino di via del Trullo, con un rilevante effetto di contenimento dei costi anche in questo settore.

un ordine del giorno chi breve ma importante per la tutela dei diritti dei lavoratori, che abbiamo già presentato lo scorso anno ma che è ancora attuale. Nasce, infatti, dalle segnalazioni fatte da alcune organizzazioni sindacali e dagli stessi lavoratori circa alcune certe inadempienze da parte delle società esterne presenti qui in Senato. È noto a tutti che è stata affidata a ditte esterne la gestione di alcuni servizi di manutenzione, pulizia, distribuzione, posta, vigilanza, informatica, e così via, nonché gli appalti per lavori di ristrutturazione dei palazzi del Senato. Come dicevo, ci sono state segnalate varie inadempienze legislative e contrattuali da parte di queste ditte nei confronti dei loro dipendenti impegnati presso il Senato: tra queste, ricordiamo i ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il mancato rispetto dell'inquadramento contrattuale e persino, signora Presidente, l'inosservanza delle norme che tutelano la maternità, oltre agli impedimenti allo svolgimento di alcune assemblee sindacali e il non riconoscimento del diritto di rappresentanza sindacale. Con questo ordine del giorno chiediamo dunque dì attuare un costante monitoraggio ai fini di un'attenta verifica del rispetto, da parte dì queste società fornitrici di servizi o titolari di appalti di lavoro della legislazione sul lavoro e delle norme dei contratti collettivi di categoria. È inaccettabile infatti, signora Presidente, onorevoli Questori, che nel palazzo in cui le leggi vengono prodotte, discusse e approvate si affidino alcuni servizi a società che non rispettano né le leggi, né i diritti basilari dei lavoratori. Con questo ordine del giorno, si intende impegnare quindi il Consiglio di Presidenza ed il Collegio dei senatori ad attuare un costante monitoraggio ai fini di un'attenta verifica del rispetto da parte di queste società fornitrici della legislazione sul lavoro e delle norme dei contratti collettivi di categoria. Confidiamo di avere questa vigile verifica e, quindi, ringrazio.

Azzollini), la spesa totale del Senato ha conosciuto una evoluzione incompatibile con lo stato della finanza pubblica e, ancora di più, con l'esigenza di un salto di qualità nella capacità della politica di guidare il Paese in uno sforzo di crescita nella stabilità; crescita nella stabilità che ci manca ormai da venti anni. Basta leggere, senatore Malan, la tabella di pagina 97 del fascicolo che contiene il bilancio. Nel 2000, la spesa totale dello Stato è ammontata a 521 miliardi,

mentre quella del Senato di 603 milioni. Ecco l'andamento incompatibile della spesa del Senato rispetto all'andamento complessivo della spesa dello Stato. Una spesa dello Stato che noi - è vero presidente Azzollini? - semmai critichiamo per un'evoluzione troppo dinamica, soprattutto per la sua componente corrente, nella fase che ci sta alle spalle. E sono 10-11 gli anni cui si fa riferimento, quindi *pro quota* attribuiamoci tranquillamente la responsabilità, ma discutiamo tra di noi, seriamente, di quello che ci dicono i numeri e dell'esigenza di porre rimedio attraverso un'azione, anche in questo campo, di riforma. Tornerò su questa tabella, perché testimonia, senatore Malan, che nell'anno in corso noi abbiamo un'evoluzione della componente della spesa del Senato

con un aumento significativo, in un contesto nel quale abbiamo, con il decreto-legge n. 98, sacrosantamente impostato una manovra che corregge nel tempo, per 47 miliardi di euro, l'andamento della finanza pubblica nel suo complesso? È chiaro che tra questi due andamenti c'è incompatibilità. Diciamocelo, perché questo è oggetto di una valutazione politica che non può non essere condivisa. Mi rifiuto di credere che non sia condivisa. Lasciate perdere la campagna di stampa, le valutazioni malevole, le considerazioni false. Lasciate perdere tutto questo. Affrontiamo ciò che ci dicono i numeri. I numeri testimoniano di un andamento della spesa totale del Senato incompatibile con le esigenze di contenimento della finanza pubblica e soprattutto con gli obiettivi, per fortuna ambiziosissimi, che abbiamo per metà di questo decennio, cioè il pareggio strutturale di bilancio. Ora, se questo è vero, allora noi abbiamo di fronte un imperativo categorico, che non riguarda il centrosinistra o il centrodestra, ma tutti noi: noi: dobbiamo recuperare nei prossimi cinque anni (si tratta di un obiettivo realistico), realistico), attraverso un crescendo di azioni riformatrici, tutto ciò che nella spesa del Senato ha ecceduto il livello coerente con il ritmo di inflazione reale di questi ultimi dieci anni. reale di questi ultimi dieci anni. Siccome abbiamo speso largamente di più di quello che sarebbe stato lecito negli anni passati, nei prossimi tre anni dobbiamo spendere molto di meno, formulando gli obiettivi in termini di spesa nominale. Come dobbiamo fare - ecco la discussione che dobbiamo sviluppare tra di noi - per conseguire questi risultati? Sono forse essi impossibili? La discussione infatti potrebbe anche concludere che non possiamo farcela, date le rigidità, che conosco bene quando si affrontano temi che riguardano un bilancio di una pubblica amministrazione. se vogliamo discutere seriamente di come si fa, dobbiamo prendere esempio dalle soluzioni adottate dai Paesi che, nel corso di questa ultima fase della storia recente, hanno affrontato problemi di riduzione significativa della spesa pubblica. Cosa hanno fatto questi Paesi? Una prima scelta fondamentale. Senatori Questori, se il Regolamento non lo consente cambiamolo tra cinque minuti, ma dobbiamo allungare risolutamente il periodo di programmazione vincolante. Non c'è nessuna possibilità di ridurre la spesa in modo significativo se decidiamo anno su anno e, addirittura, anno

bilancio pluriennale vincolante, che ogni anno viene modificato in base all'andamento delle cose reali: ma l'obiettivo deve essere formulato in termini pluriennali e crescenti. Se ci sono almeno cinque anni di programmazione, allora i vincoli si allentano e tutto diventa più facile. Se non ci sono, tutto è impossibile. Questa è la prima indicazione metodologica. La seconda nasce di conseguenza: bisogna avviare immediatamente una scientifica - sissignori: scientifica revisione totale della spesa adottando il metodo del bilancio a base zero. Ogni euro deve essere giustificato dall'inizio. Nessuna spesa deve essere fatta domani per la sola ragione che l'abbiamo fatta sempre e in particolare ieri: nessuna

Quindi, nell'ambito di questa radicale revisione della spesa, feroce fino all'ultimo euro, che rigiustifica tutto, dal primo euro di spesa fino all'ultimo, è chiaro che bisogna scegliere di concentrarsi sul *core business*: legislazione e controllo.

Se assumiamo questo insieme di obiettivi in termini nominali, recuperiamo quello che abbiamo speso per responsabilità di tutti (volete che dica prima di tutto la mia? Benissimo: prima di tutto la mia) negli anni scorsi più di quello che potevamo e dovevamo spendere. Quarto: lungo quali indirizzi? L'indirizzo è chiaro: ci sono spese che si giustificano con la specificità del Senato, quelle devono essere affrontate con specifiche appostazioni, che hanno una loro logica ed evoluzione. Poi c'è il resto della spesa. Per esempio, il trattamento previdenziale dei dipendenti. Qualcuno si è chiesto perché non diciamo quello che noi spendiamo per il trattamento previdenziale dei dipendenti? Ve lo dico io perché: perché se non avessimo un sistema interno dovremmo avere i dipendenti nell'ambito del sistema INPS o INPDAP; ma allora i contributi sarebbero diversi, il calcolo della prestazione sarebbe profondamente diverso. Io qui sono per adottare un criterio che dice che per i dipendenti il metodo di calcolo, il metodo di contribuzione, la dimensione della contribuzione, la dimensione delle prestazioni sono adottati secondo la logica del sistema previdenziale di tutti i comuni mortali, per il Senato, per la Camera, per la Presidenza della Repubblica e per la Corte costituzionale. Naturalmente questo implica che anche per il nostro vitalizio si adotti il metodo di calcolo contributivo. È ampiamente possibile farlo. Già anni fa, persino quando feci la relazione io, senatore Malan, riuscii a proporre questo (se lei va a vedere gli atti controllerà la naturalmente nessuno «mi si filò», come sempre in questi casi. Tuttavia, la proposta è ovvia: adottiamo per il nostro vitalizio il metodo di calcolo che si adotta per i comuni mortali. la tabella di pagina 97 dice che l'obiettivo della riduzione dell'1 per cento della nostra spesa nel 2011 è facilmente raggiungibile. Certo, ci vuole un impegno specifico per i mesi che restano, ma è un obiettivo raggiungibile, che io considero di cruciale rilievo, non per andare in giro a dire che

quello che spendiamo nel permanente, evidentemente non andiamo da nessuna parte nel conseguire gli obiettivi che proponiamo che il Senato si dia. Su questa base, è possibile un dialogo tra di noi? Non tra maggioranza e opposizione, ma tra senatori che vedono che c'è una crescente contestazione nel Paese, non solo sulla base degli articoli dei giornali o delle comunicazioni televisive, e così via (che hanno tutti i vizi che conosciamo), sulla base della considerazione di dati di fatto. L'altro giorno alla Camera dei deputati - mi verrebbe voglia di predisporre un ordine del giorno per dire esplicitamente di non applicare quell'accordo - hanno giustificato l'aumento dell'indennità fissa dei dipendenti

Ma, signora Presidente, lei sa cosa prevede quell'accordo straordinario sull'assenteismo? Prevede che se per caso quest'anno vengo a lavorare sempre e non faccio assenze ingiustificate per malattie inesistenti, il prossimo anno sto a casa cinque giorni! Ma siamo matti? Ma vogliamo andare in giro a dire che noi stiamo facendo un'operazione di risanamento perché facciamo cose di questo tipo, o vogliamo dire che ci siamo resi conto dello stato di emergenza in cui operiamo e vogliamo cambiare totalmente aria? La proposta contenuta nell'ordine del giorno del Partito Democratico è questa. Non è polemica verso nessuno; è critica verso noi stessi, quindi necessariamente autocritica, e impegnativa per tutti.

al primo punto dell'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani sarà anticipato l'esame del decreto-legge in materia di immigrazione.

ha parlato di «previe intercorse tra i Gruppi». Siccome non mi risulta che l'intesa sia stata previa, noi sosteniamo che invece sarebbe meglio

soltanto per dire che non vi sono obiezioni da parte nostra all'ordine indicato dal senatore Ferrara, nel senso che, per

ritiro la riserva, perché ritengo che così a questo punto debba essere. Ho comunque una riserva che ci possa essere stata una comunicazione non perfetta, perché la normale gestione